era una dichiarazione che facevamo preventivamente, ma non avevamo esattamente capito in che cosa potessero consistere i grandi cambiamenti che la crisi avrebbe portato. I provvedimenti che oggi arrivano alla nostra attenzione sono una prima esplicitazione di come sta cambiando il mondo dopo la crisi o, per lo meno, dopo le prime fasi della crisi. Questa, di fatto, è la seconda manovra di profondo

poiché è risultato evidente che avevamo regole che consentivano alle autorità di vigilanza (mi riferisco, in particolare, all'Europa) di vigilare all'interno dei confini dei propri Stati su soggetti che, invece, operavano *cross border*; vi erano, quindi, limiti oggettivi alla loro vigilanza. Dall'altra parte, vi sono stati errori errori di valutazione, in particolare per l'Europa, rispetto alla capacità di tenuta del Patto di stabilità europeo come strumento preventivo delle crisi di *default* degli Stati sovrani. Agli errori di vigilanza si è posto rimedio individuando degli strumenti di vigilanza vigilanza europea che tengono conto degli insegnamenti della crisi. Ci auguriamo che funzioneranno come preventivo per le prossime situazioni che non possiamo escludere si verificheranno. Per quanto riguarda, invece, la riforma per ridurre il rischio di squilibri in grado di condurre il fallimento sovrano all'interno degli Stati, questi - i provvedimenti che sono alla nostra attenzione - costituiscono, di fatto, la risposta

Solo nel gennaio di questo anno ci si è accorti di un fatto che poteva essere prevedibile, ossia che l'impatto della crisi in Europa è avvenuto in modo totalmente diverso a seconda dei singoli Stati perché è stato un impatto drammaticamente amplificato dalle vulnerabilità preesistenti. E per la prima volta ci si è resi conto che gli strumenti che erano a disposizione per valutare, per quanto concerne le situazioni degli Stati membri dell'Europa, quale fosse il loro reale stato economico e finanziario, erano strumenti impropri ed inadeguati perché, comunque, basati su parametri che si sono rivelati del tutto fallaci. perché con il Patto di stabilità la sorveglianza sulle situazioni dei singoli Stati c'è stata, ma è stata una sorveglianza che ha tenuto conto di dati numerici e non ha valutato un cambiamento sostanzialmente che era intervenuto nel frattempo, ossia che il dato numerico non bastava più. La Grecia, nel gennaio scorso, è

che dovrebbe riuscire - mi auguro - a superare i limiti che questa unione monetaria ha mostrato nell'attuale contingenza drammatica, essendo priva di un bilancio generale in grado di affrontare gli *shock* asimmetrici che si sono verificati. verificati. Questa manovra di *governance*, a mio parere, rappresenta una positività indubbia. È cioè un impianto che cambia radicalmente gli strumenti per affrontare

pianificazione di una serie di strumenti che dovrebbero essere in grado di farci affrontare in modo diverso possibili crisi che nessuno può nessuno può escludere possano ripetersi perché siamo comunque, rispetto alle crisi, internazionali, in una situazione del tutto nuova ed ancora molto difficile da decodificare. Quali rischi leggo all'interno della proposta che ci viene sottoposta? Il rischio è che si ripetano i due errori fondamentali del Patto di stabilità, che pure conteneva aspetti fortemente positivi, la certezza delle regole e la certezza delle sanzioni. Il Patto di stabilità sanciva una certezza di regole che non sono state rispettate, a partire dagli Stati potenti all'interno dell'Unione europea:

stabilità, che hanno portato sostanzialmente a maneggi di carte e a patteggiamenti che hanno reso la pena - come si dice anche in questo caso - del tutto ininfluente e la sanzione del tutto inutile. Quindi, se

come sistema europeo.

Per non parlare di cose di casa nostra, parliamo della *cagnotte* francese che, quando si è realizzata, è stata regolarmente redistribuita e non è certamente andata ad un miglioramento dei conti generali. generali. Credo che un'ulteriore necessità, su cui mi auguro che il Governo riesca in sede europea ad ottenere risposte positive, sia quella di creare un soggetto autonomo

sempre detti - alla possibilità di adattamento della nostra economia, particolarmente in caso di *shock* che possono avere avere conseguenze irreversibili. Un secondo *shock* oggettivamente sarebbe molto difficile da reggere per il nostro Paese. È stato giustamente sottolineato il fatto, cui assegno una forte valenza, che

solo una volta e non può ripetersi, perché i risparmi che le generazioni precedenti hanno accumulato anziché spendere non si spendono due volte. Quindi, in caso di un secondo *shock*, non avremo più il grande materasso che ha attenuato questa crisi.

L'Istituto Bruno Leoni ha fatto una cosa interessante: l'orologio del debito. Mi auguro che venga installato con l'aiuto di noi tutti per rendere il debito evidente fisicamente all'esterno, a tutti, perché ci sia una consapevolezza collettiva. Parlare di debito è questione che in Aula torna spesso e nella testa della gente è cosa molto lontana, invece le conseguenze di questo debito saranno nei prossimi anni - lo ha ricordato bene il senatore Giaretta - molto pesanti sulle spalle di tutti. È bene allora che cominci ad esserci una consapevolezza collettiva di quale sia il debito di questo Paese, di quali sono le conseguenze che il debito porta e, quindi, di quali siano le politiche ineludibili per superarlo.

1.640.000 euro. In questi 10 minuti, 1.640.000 euro in più è quanto si sta aggiungendo nel debito pubblico. questo numero sia sufficiente per far sentire sulle nostre spalle la responsabilità forte che abbiamo come istituzioni nei confronti di questo problema e della sua soluzione. Reputo estremamente positiva, all'interno della Commissione bilancio, in ordine a questi strumenti che si stanno approntando a livello europeo (e che sicuramente creeranno sicuramente creeranno anche pressione all'interno del nostro Paese) perché si vada rapidamente nella direzione della riduzione del debito, l'unanimità sostanziale intorno al provvedimento, che depone a favore di una consapevolezza diffusa della necessità della necessità di non sottovalutare questo problema e di non attendere tempi diversi per affrontarlo.

ci imporranno di rientrare e lo faranno in tempi decisamente brevi e con oneri decisamente forti. Questo allora significa che c'è un rischio forte di scardinare l'ossatura del Paese, le sue certezze e i suoi standard di vita. Da ciò, di cui oggi stiamo discutendo, in termini talvolta anche un po' accademici, esce una trasformazione del Paese, di cui facciamo fatica in questo momento a renderci conto. Certo, la trasformazione potrà avere facce totalmente diverse a seconda degli approcci e dei programmi che si faranno. Per questo, è bene che si arrivi in fretta alla proposta che gli atti di oggi sottengono, ossia come il nostro Paese rientra da questo debito, come

andremo incontro sicuramente ad un sovraccarico delle competenze, delle prerogative, delle funzioni che il Parlamento dovrà svolgere, perché dovremo tornare a discutere degli schemi di regolamento della Commissione e del Consiglio riguardo a tutta la politica di sorveglianza dei bilanci pubblici

come si pensa o si vuol far credere, che il nuovo Patto di stabilità e crescita, che dovremo presentare all'Europa prima del 15 aprile, non sia altro che una sorta di fotocopia rispetto a quello che il Parlamento italiano già faceva con la relazione unificata di economia e finanza. Dovremo continuare a discutere - e lo faremo a breve - del Programma nazionale delle riforme; anche in questo caso, l'Europa ci chiede, attraverso questo Programma nazionale, nazionale, degli impegni precisi. Non è un elenco della spesa, un libro dei sogni, una sommatoria di annunci o di proclami, si tratta di un piano di riforme che debbono avere una loro specifica validità; così come il Patto di stabilità e crescita che l'Europa ci chiederà non è semplicemente un un annuncio di stabilizzazione di conti pubblici, ma si tratta di programmi di politiche di bilancio a medio termine che devono avere precisi riscontri.

Oggi e domani, il 28 e 29 ottobre, il Consiglio europeo è stato chiamato a discutere sia dei punti controversi del rapporto del rapporto della *task force*, sia degli orientamenti che i singoli Stati membri vorranno dare a questo rapporto. Non c'è nulla di deciso, non c'è nulla di definito. Oggi la stampa nazionale e internazionale riporta che le posizioni tra la Commissione e il Consiglio europeo sono ancora

Innanzitutto il problema del debito pubblico, che è stato abbondantemente ricordato in quest'Aula. Chiunque di voi ha avuto modo di leggere esattamente i contenuti delle proposte che provengono dalla Commissione dal Consiglio si è reso conto che tra i vari schemi vi sono posizioni per affrontare il debito pubblico completamente differenti tra loro. Da un lato c'è il meccanicismo nel processo di risanamento del debito pubblico: questo comporterebbe per il nostro Paese - lo abbiamo detto più volte - manovre finanziarie dell'ordine di 3 o 4 punti di PIL annuali, con importi dell'ordine di 30 o 40 miliardi di euro; dall'altro lato, vi è una proposta di sostenibilità del debito pubblico attraverso un insieme di indicatori. Occorre

si è affrontata la possibilità di parlare di debito aggregato (quindi non solo di quello pubblico, ma anche di quello privato). Non è così, Non è così, perché, considerando la sostenibilità del debito pubblico nella sua formulazione più confacente per il nostro Paese, comunque noi,

nel 2013-2014 avanzi primari dell'ordine del 3-3,5 per cento. Ci rendiamo allora conto di come gli impegni del nostro Paese siano particolarmente stringenti in questo senso. senso. Il secondo punto che il rapporto della *task* *force* ha messo in risalto è la verifica e la decisione in merito agli indicatori di sorveglianza.

non sono solo indicatori di rischio di bilancio, come possono essere le scadenze o lo *stock* del debito pubblico. Sappiamo anche che oltre metà del debito pubblico nel nostro Paese è in mano a investitori esterni, a investitori stranieri, i quali giudicano la credibilità del nostro Paese

Ecco perché dovremo ragionare anche sugli altri indicatori di sorveglianza che sono estremamente importanti e che l'Europa ci ha chiesto di esaminare. Il primo indicatore è l'aggiustamento della spesa. Lo dico al Governo, che si era fatto portabandiera della salubrità dei conti pubblici. Abbiamo chiuso il 2009 con un aumento della spesa primaria corrente una riduzione della spesa in conto capitale per gli investimenti. È previsto, in base alla Decisione di finanza pubblica, un leggero miglioramento in termini di riduzione della spesa pubblica nei prossimi due anni, e di nuovo un aumento nel 2013. Ci rendiamo allora conto che l'aggiustamento della spesa pubblica non potrà avvenire come è stato fatto finora, con tagli lineari, con tagli che falcidiano i settori più importanti del nostro Paese: la scuola, la ricerca, l'innovazione.

facendo parte del sistema dell'Unione europea, non potrà incidere attraverso una svalutazione dell'euro o una riduzione dei prezzi o dei salari, tal modo non produrremo altro che deflazione e recessione: dovremo agire inevitabilmente sulla produttività del nostro sistema Paese. E le riforme che ci attendono non potranno avere efficacia il giorno prima per il giorno dopo: pertanto, oggi, e non domani, dobbiamo cominciare ad agire. Ecco perché il Piano nazionale di riforma, che l'opposizione ha voluto fosse oggetto

scoperto. Ha fatto bene il presidente dell'Eurogruppo Juncker a dire che il diavolo sta nei dettagli che devono essere ancora scritti.

*(PD)*. Signor Presidente, questa mattina i principali quotidiani europei riferiscono del dibattito in corso e delle problematiche politiche, istituzionali ed economiche che la riforma della *governance* economica europea, di cui stiamo discutendo,

Sarkozy, e sulla necessità di modifica dei trattati in modo tale che le sanzioni e le regole in via di definizione siano più incisive, fino a prevedere la sospensione del diritto di voto per i Paesi inadempienti alle regole che si stanno costruendo. Andiamo in Italia, invece. La discussione che stiamo facendo al Senato e che non si sta facendo alla Camera dei deputati dei deputati è stata, come è a tutti noto, determinata da una precisa richiesta dell'opposizione e, in particolare, del nostro Gruppo. La discussione si sta svolgendo in una disattenzione abbastanza estesa anche in questo ramo del Parlamento, certamente nella disattenzione del Governo (ringrazio il sottosegretario Casero qui presente, ma mi sembra che il Governo ai suoi massimi livelli sia impegnato in altre faccende) e, soprattutto, nella disattenzione dei *media*. Eppure, come è stato detto da tutti i colleghi intervenuti, stiamo discutendo di nuove regole nei rapporti tra l'Unione europea e gli Stati membri destinate ad incidere profondamente non soltanto nei rapporti comunitari all'interno dell'Unione europea, ma sulle decisioni di bilancio nazionali, sulla tempistica dei documenti di bilancio, sui contenuti dei documenti di bilancio, sul programma delle riforme strutturali che saranno necessarie per rispettare i nuovi obiettivi che si decideranno in Europa nonché sul tema, decisivo per la vita del del nostro Paese, del coordinamento di un programma di riforme credibili con una nuova politica di bilancio. Questi programmi incideranno profondamente su ciò che dobbiamo decidere nei prossimi giorni, settimane, mesi fino ai prossimi venti anni almeno, in particolare per le modalità e l'entità della riduzione dell'enorme debito pubblico che abbiamo accumulato nel corso dei decenni. dibattito coinvolge l'Europa e i 27 Paesi membri; coinvolge tutti, ma se c'è un Paese che dovrebbe prestare più attenzione degli altri, dovrebbe interrogarsi di più e assumere decisioni più forti e incisive è il nostro, contrariamente a ciò che sta avvenendo per le ragioni che tutti conosciamo e di cui abbiamo ampiamente dibattuto in questi anni. Mi riferisco all'altissimo livello del debito, alla rigidità nella composizione della spesa pubblica, che rende per lo più inefficaci gli interventi di correzione che sono stati decisi e adottati nel corso del tempo, al livello record della spesa e della pressione fiscale e, quindi, ai margini ristrettissimi che abbiamo nella manovrabilità del bilancio pubblico che hanno imposto, impongono e imporranno decisioni dolorose per gli squilibri macroeconomici enormi di cui si è discusso è discusso e che esistono, per il basso tasso di crescita, per la costante riduzione del livello di competitività che registriamo da molti anni a questa parte. Vi sono moltissime ragioni che che indurrebbero il nostro Paese, non solo ad essere più attento e più presente in questo dibattito, ma a capeggiare ed essere tra i protagonisti di questo confronto in Italia e in Europa. Nel merito, signor Presidente, non saprei dire di più e meglio di quanto hanno detto i colleghi del gruppo del Partito Democratico che sono intervenuti e che interverranno. D'altronde, siamo agli inizi di questa discussione: avremo tempo per approfondirne i vari aspetti poiché i contenuti di questo percorso e di questa discussione ci occuperanno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e, quindi, torneremo sul merito di molte delle problematiche che verranno sintetizzate nelle decisioni che gli organismi comunitari si apprestano ad adottare. Voglio invece proporre qualche riflessione su come il nostro Paese arriva a questo appuntamento storico ed importante, a questo passaggio epocale sotto l'aspetto della gestione delle politiche di bilancio, non per le sue condizioni finanziarie o economiche - che ci sono note

non per alimentare polemiche politiche, che abbiamo già svolto a tempo debito e che, nel caso, saremo costretti a riproporre, ma per tentare di fornire un metro di misura dell'enorme distanza che ci separa

primo luogo, come è stata gestita la politica di bilancio ed economica in questi due anni e mezzo? Il grosso delle decisioni

della sessione di bilancio, a cui sono seguite leggi finanziarie o di stabilità vuote, senza alcuna visione senza alcun disegno di riforma che accompagnasse gli interventi finanziari correttivi e con un ruolo del Parlamento nazionale che è risultato vieppiù marginale.

economica, ponendo il dibattito ed il confronto parlamentare al centro delle decisioni. Si è verificato un accentramento sostanziale di tutte le decisioni in questa importantissima

in occasione dell'esame della Decisione di finanza pubblica, leggendo le note del Servizio del bilancio e i documenti che abbiamo esaminato, ho contato otto violazioni della legge di contabilità in tre mesi: in tre mesi: il 15 luglio dovevano essere presentate le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica e non sono state presentate (adempimento totalmente omesso); il 15 settembre doveva essere presentata la Decisione, che invece è stata presentata il 30 settembre; è stata omessa l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio, il cosiddetto scenario macroeconomico a politiche invariate (peraltro, questo problema si ripresenterà perché il decreto-legge che il Governo sta preparando dovrà affrontare il tema delle risorse necessarie per confermare gli impegni assunti). Inoltre, in quel documento manca l'indicazione dell'obiettivo della pressione fiscale massima,

auspichiamo, dovrà ridursi); non vi sono indicazioni sul contenuto del Patto di stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali (anche questo è un tema cruciale, previsto nella legge di contabilità); non sono state allegate le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa e le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali; manca il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale; infine, si è verificata quella enorme violazione, che abbiamo qui denunciato

questione dei fabbisogni standard è stata affrontata con un decreto vuoto, che rinvia ad un provvedimento amministrativo successivo, con un percorso che non contempla alcun disegno di coordinamento della finanza locale e territoriale con la politica di bilancio nazionale. Infatti, non vi è traccia degli effetti finanziari oltre che ordinamentali del federalismo fiscale nei documenti di bilancio dell'anno prossimo e del prossimo triennio. Ma il federalismo non doveva essere, dal vostro punto di vista ma anche dal nostro, seppure partendo da idee e presupposti differenti, l'avvio differenti, l'avvio di un percorso virtuoso per la riduzione della spesa e del debito? Quante volte abbiamo sentito questa affermazione nelle Aule parlamentari e nel dibattito pubblico? Eppure, nella fase

tra i vari territori. Facciamo ancora in tempo a correggere questa rotta, purché la maggioranza decida di smettere di fare propaganda su tale tema e di collocare l'attuazione seria e rigorosa

rilevante sulle decisioni che dovremo assumere nel prossimo futuro. che la discussione, che noi abbiamo chiesto e voi avete accettato di svolgere, si concluda con una risoluzione unitaria. È un fatto assolutamente positivo, e mi sento di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, a partire dal presidente Azzollini, e poi tutti i componenti della Commissione bilancio,

procedurale, di ripristino di un corretto rapporto tra Governo e Parlamento nel prossimo futuro, se vogliamo dare corso agli impegni contenuti nella risoluzione, e soprattutto metterci in linea in linea con le indicazioni che verranno dalla riforma in sede comunitaria, dovremmo fare l'esatto contrario di quanto avete fatto in questi due anni e mezzo nella gestione delle politiche di bilancio e nella ideazione,

per il bene e nell'interesse del Paese, di sbagliarmi. Credo però che questo Governo e la sua maggioranza non abbiano la determinazione e la forza per poter cambiare radicalmente il modo di approcciare queste problematiche, ripristinando in primo luogo il corretto rapporto tra Governo e Parlamento. Ciò che è certo è che da subito invece il nostro Paese e il nostro Parlamento hanno la necessità di cambiare passo e direzione.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, intervengo non a nome del mio Gruppo ma per mandato dalla 14a Commissione del Senato, la quale mi ha incaricato di questo nella seduta della Commissione di ieri pomeriggio. L'Assemblea del Senato si trova oggi a discutere un argomento cruciale per il futuro dell'Unione europea e del nostro Paese, ossia la nuova *governance* europea, allo scopo di trasmettere al Governo alcune proposte di indirizzo per l'imminente riunione del Consiglio dell'Unione europea. L'auspicio della 14a Commissione è naturalmente che la nostra Assemblea sia sempre più coinvolta nel dibattito delle questioni europee. Siamo convinti della necessità di aggiornare i criteri della *governance* europea, criteri che ci permettano di superare in modo migliore momenti di crisi, ma soprattutto di prevenire situazioni come quella che abbiamo recentemente vissuto e che già altri colleghi hanno ricordato. Questo tema è all'attenzione di tutte le istituzioni europee. Anche l'altro ieri, nella riunione plenaria delle Commissioni specializzate negli affari europei dei 27 Paesi dell'Unione, il presidente della Consiglio europeo Van Rompuy si sono soffermati a lungo su di esso. Soprattutto il presidente Van Rompuy ha illustrato all'assemblea della COSAC le conclusioni della *task force* creata appositamente. Non è un segreto che la posizione della Commissione è diversa dalle conclusioni della *task force*: più rigida la posizione della Commissione, che non vuole cedere sull'introduzione di *target* numerici di riduzione del debito, più flessibile quella della *task force* nell'ottica di una riforma della *governance* economica non solo punitiva, ma che induca i Paesi a ridurre i deficit di bilancio in modo proporzionale rispetto alla crescita, che tenga conto di indicatori macroeconomici e dell'efficienza dei Paesi più in generale. Questo, per non bloccare definitivamente, in un momento così difficile per la ripresa, la possibilità di sviluppo. Nel merito delle procedure - e mi soffermo sul merito, perché spesso esso è anche sostanza - penso che vada però fatta qualche precisazione.

Ciò che mi preme però evidenziare è che i Parlamenti nazionali hanno otto settimane per esprimere i loro pareri su questi documenti che ci ha inviato la Commissione e che, a norma di regolamento, il Consiglio non potrebbe in nessun modo chiudere l'esame del dossier senza aver ricevuto i suddetti pareri e del Parlamento europeo. Ricordo che il Parlamento europeo, codecisore sull'argomento, è ben lontano da una qualsiasi presa di posizione su questo punto addirittura non è stato ancora nominato il relatore. Tengo quindi a precisare che, pur ritenendo molto utile, importante, fondamentale aggiungere tutti gli aggettivi che riteniamo e che abbiamo già ascoltato in quest'Aula - il dibattito odierno in vista di una scadenza molto prossima (la prima è quella del prossimo Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre e l'altra è quella del 12 novembre) deve essere assolutamente chiaro che qualunque risoluzione venga approvata oggi non può precludere, in alcun modo, l'esame dettagliato delle proposte che la Commissione ci ha inviato,

Signor Presidente, meno di due mesi fa, lo scorso 1° settembre, sulle colonne de «Il Sole 24 Ore» e del «Washington Post» Charles Kupchan, definito dal presidente Napolitano un valoroso osservatore americano non ostile all'Europa, scriveva che «l'Unione Europea sta morendo». «Il declino dell'Europa» - scriveva Kupchan - «in parte è economico. La crisi finanziaria ha colpito duramente molti stati membri, e i livelli del debito pubblico e la salute incerta delle banche del continente potrebbero essere presagio di altri problemi in futuro. Ma sono malanni di poco conto in confronto ad una malattia più seria: da Londra a Berlino e a Varsavia, l'Europa sta assistendo a una rinazionalizzazione della vita politica, con gli stati che fanno di tutto per riprendersi quella sovranità che un tempo erano disposti a sacrificare per l'obiettivo di un ideale collettivo». Le parole di Kupchan sono quelle di un innamorato deluso. Solo pochi anni fa, l'ex consigliere di Clinton aveva scritto un libro per sostenere la tesi che se il XX era stato il secolo americano, il XXI sarebbe stato il secolo europeo. E invece, dinanzi alla prova dura della crisi economica, l'Europa ha vacillato e in particolare la crisi greca ha gettato scompiglio nelle barocche regole dell'Unione, con gli Stati membri che sono parsi, a tratti, reagire come un formicaio impazzito tra "si salvi chi può" e "tutti contro tutti".

Napolitano sapeva che due giorni dopo, il 6 e il 7 settembre, i Ministri finanziari dell'Unione si sarebbero riuniti a Bruxelles in un vertice straordinario per riscrivere, nell'ambito della *task force* guidata dal presidente Van Rompuy, il Patto di stabilità e crescita, cioè la costituzione finanziaria ed economica dell'Unione. Proprio stamani il Consiglio europeo sta decidendo sulle proposte della *task force*, che in gran parte la Commissione ha già tradotto in proposte di legislazione secondaria. Sapremo nelle prossime ore se quella di oggi sarà una giornata storica per l'Europa. Quel che è certo è che con il pacchetto elaborato dalla *task force* l'Europa, data per morta, non solo tenta di rialzarsi, ma prova a fare un salto di qualità nel processo d'integrazione. Come osservava il 5 settembre scorso Giuliano Amato, anche lui rispondendo a Kupchan (riassumo la sostanza del suo ragionamento), dal Trattato di Maastricht fino ad oggi, da quando cioè decidemmo che le politiche economiche e finanziarie rivestivano un interesse comune, ci siamo dati regole che rendessero le politiche nazionali compatibili con alcuni standard comuni. La crisi ci ha imposto e ci sta imponendo un salto di qualità. È diventato improvvisamente ineludibile produrre ciò che mai era stato chiesto ai leader dei Paesi europei di produrre: non più solo il coordinamento europeo di politiche nazionali, ma politiche economiche sia sul versante della finanza pubblica sia su quello macroeconomico dell'economia reale, politiche davvero europee. La proposta di semestre europeo contenuta nel pacchetto della *task force* è da questo punto di vista clamorosa: dal 2011 non solo la manovra di bilancio ma le stesse riforme economiche e sociali non saranno più strumenti nazionali da fare rientrare entro parametri comuni, ma la traduzione nazionale, rigorosamente controllata e verificata, di decisioni europee. Insomma, sta succedendo, potrebbe succedere, l'esatto contrario di quel che teme Kupchan. Pure in un contesto di evidente rinascita dei nazionalismi, non solo gli Stati non si riprendono la loro sovranità magari vorrebbero farlo ma non ci riescono -, ma ne cedono all'Unione un'altra quota e una quota assai significativa. Come sempre accade per l'Europa, ogni progresso apre nuovi problemi e pone nuove sfide. La prima sfida sarà nello stesso nuovo Patto di stabilità e di crescita. Qualunque sia il livello di durezza delle sanzioni, difficilmente avrà successo la politica europea di stabilità senza contemporaneamente una politica europea di sviluppo. Il rilancio della proposta Delors, contenuta nel Libro bianco del 1992, di istituire un fondo europeo per grandi investimenti, finanziato attraverso *eurobond*, dal nostro punto di vista sappiamo essere largamente condiviso nel nostro Paese a cominciare dal ministro Tremonti - è uno strumento di vitale importanza. Poi c'è il tema dell'architettura istituzionale. Non a caso, polemiche quotidiane a parte, Angela Merkel e Nicholas Sarkozy hanno cominciato a parlare di revisione dei Trattati. il Trattato di Lisbona, che pure ci è costato sudore e brividi, più di una salita di sesto grado, è già superato dalla storia, che è andata più avanti. Se la sovranità della politica economica si sposta dagli Stati membri all'Unione, dobbiamo decidere chi la esercita. Se la costituzione formale dell'Europa resta quella attuale, la sovranità sarà esercitata da un concerto di Stati diretto dallo Stato più forte, che oggi è la Germania: ci piaccia o no, la capitale d'Europa sarà, anzi, per molti versi già lo è, Berlino. Se vogliamo che resti a Bruxelles, dobbiamo dare all'Europa non uno Stato - l'Europa è costitutivamente poliarchica - ma un Governo e un Presidente eletti dai popoli e bilanciati dagli Stati e dal Parlamento. Questa è la nuova sfida che l'Europa ha davanti a sé, che noi europei abbiamo davanti a noi. La seconda sfida, signor Presidente, riguarda noi italiani; purtroppo è una sfida, diciamo così, meno aulica. Fino a quando il Governo europeo sarà la riunione dei Governi, l'unica legittimazione democratica delle decisioni europee resta per ora quella dei Governi nazionali. Questo dato di fatto rende incompatibile con la democrazia una gestione opaca del circuito tra proposte nazionali e decisioni europee, come quello che si è registrato in modo clamoroso e scandaloso in questo passaggio storico. Complice un'opinione pubblica che il sistema dei *media* sta affogando nella stupidità, nel populismo di destra e di sinistra, facendo largo e abile uso delle armi di distrazione di massa - basta sfogliare i giornali di oggi il Parlamento e le forze politiche sembrano non essersi quasi accorti del passaggio epocale che stiamo vivendo. Ma il Governo, sia quello politico, benché di fatto in crisi da mesi, sia quello tecnico (di cui parlava ieri il collega Morando), il Governo monocratico del Ministro dell'economia, che da mesi agisce e decide in solitudine, non può pensare di avere - in un passaggio come questo - una delega in bianco che lo esenti perfino dal rispondere al Parlamento delle proposte avanzate e delle linee di condotta tenute in sede europea. Ieri sera abbiamo visto il ministro Tremonti cenare al ristorante del Senato: avremmo preferito vederlo in Aula, magari insieme al Presidente del Consiglio, che formalmente ci dicono sia ancora in carica. Sarebbe stato interessante e forse utile al Paese, certamente rispettoso della forma e della sostanza della democrazia, che avessero riferito al Parlamento, il primo, del lavoro fatto in seno alla *task* *force* abbiamo dovuto apprendere in questi giorni dai bollettini europei di un contributo scritto dall'Italia alla *task force* e depositato nel mese di luglio, del quale il Parlamento non ha mai saputo nulla e il secondo, il Presidente del Consiglio, degli orientamenti che avrebbe sostenuto oggi, che sosterrà oggi. Cosa pensa il Presidente del Consiglio della riforma dei Trattati di cui stanno discutendo il Cancelliere tedesco e il Presidente francese in seno al Consiglio europeo? Il Partito Democratico ha chiesto e ottenuto questo passaggio parlamentare, ma il Governo, ancora una volta, ha scelto di sottrarsi al confronto: basta guardare la desolazione di quei banchi. Lo rileviamo con rammarico e preoccupazione. Noi lavoreremo per costringerlo a cambiare linea di condotta: ne va della democrazia nel nostro Paese, del ruolo del Parlamento e della capacità del popolo italiano di essere rappresentato adeguatamente in Europa.

rispetto alla pur alta qualità del dibattito che si è svolto in quest'Aula, oltre che in Commissione, in questi giorni. giorni. È all'esame di questa Assemblea la risoluzione sulle procedure di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche europee che costituiscono, senatore Tonini, l'espressione di un indirizzo

e che probabilmente - e vengo ad alcune delle sue osservazioni, senatore Tonini - affiderà proprio a quella *task force* che lei ha citato opportunamente il mandato, addirittura, per esplorare possibilità e necessità di procedere alla modifica del Trattato di Lisbona. Risoluzione costruita sulla scorta di documenti tecnici, quelle proposte di regolamento e di direttiva approvati dalla Commissione il 29 settembre scorso; documenti ampiamente esposti dal relatore e dagli intervenuti nel corso della discussione, sia in Commissione che qui in Aula, che danno conto del quadro della nuova e complessa normativa che va delineandosi in materia di *governance* economica comunitaria. Criteri che nascono dalle criticità e dalle emergenze messe in evidenza dalla crisi, che intendono rafforzare la *governance* stessa e porre al riparo l'integrazione economica e finanziaria raggiunta dall'UE da possibili future difficoltà. ancora, probabilmente, ne dovremo ancora affrontare. Cambiamenti sostanziali, in ordine alla necessità di definire strumenti regolatori, meccanismi di gestione e poteri sanzionatori, più volte richiamati anche dall'intervento della senatrice Leddi. Da un lato, quindi, le nuove regole agiscono per introdurre una maggiore cogenza nell'applicazione della disciplina di bilancio prevista dal Patto di stabilità e crescita, confermandone tuttavia la sostanziale validità, così come ha ben sottolineato il senatore Morando nei suoi interventi sia in Commissione che in Aula. Regole fondate sul concetto di rigore e sostenibilità delle finanze pubbliche, premessa assolutamente indispensabile per qualsiasi politica di sviluppo e di crescita. Non a caso, gli interventi previsti per la componente preventiva del Patto si basano su un controllo delle finanze pubbliche fondato sulla prudenza, coniugato alla convergenza a medio termine verso il pareggio di bilancio. Così come nella parte correttiva del Patto al meccanismo di monitoraggio e di rientro del deficit, già previsto all'interno delle procedure per i disavanzi eccessivi, viene affiancato un analogo procedimento per il debito e il suo rapporto con il PIL dal quale, certo, non potremo prescindere. Del resto, quelle regole tendono alla creazione di una rinnovata e più forte sorveglianza macroeconomica sugli squilibri di competitività e crescita, basata su una serie di indicatori economici "non convenzionali", tra cui il debito di famiglie e imprese, le partite correnti, il costo del lavoro. In sintesi, un sistema di sorveglianza macroeconomica che diventa complementare agli interventi migliorativi sul Patto di stabilità e crescita e sul quale si gioca, in fondo, la partita. Regole, non dobbiamo dimenticare, che vanno ad affiancarsi a quel meccanismo *ex ante* di coordinamento delle politiche economiche, quelle contenute nel cosiddetto semestre europeo, già operativo a partire dal prossimo gennaio, volte a rafforzare la disciplina di bilancio e la stabilità macroeconomica. Una questione molto importante e molto ben evidenziata nella sua difficoltà applicativa per il nostro Paese con le perplessità già espresse dal relatore. Ieri, come è stato ricordato, in visita al Senato c'era la Corte dei conti europea. Ringrazio la presidente Boldi per aver voluto dare l'opportunità agli Uffici di presidenza della Commissione e alle Commissioni competenti e interessate l'opportunità di confrontare con i membri della Corte dei conti europea anche questi temi, anche queste questioni così profonde relative al controllo e alla verifica dei conti europei, non solo in ordine all'utilizzo dei fondi strutturali ma proprio a quelle politiche di coordinamento. proposta di risoluzione all'esame di quest'Aula non può non tener conto delle conclusioni cui è già pervenuta una decina di giorni fa la *task force* sulla *governance* economica del Consiglio europeo, ossia di quel documento politico che interviene nel segno della flessibilità su alcune proposte della Commissione: un documento «senza numeri» - come lo ha definito il ministro Tremonti - che costituisce invece, senatore Tonini, per chiarire alcune sue perplessità, un significativo passo avanti verso la definizione di una *governance* economica dell'Unione europea; una sintesi delle diverse impostazioni ed aspirazioni nazionali, basata sulla logica di apportare cambiamenti sostanziali alla stessa *governance* in riferimento al livello di integrazione economico-finanziaria raggiunta, tenendo conto tuttavia della necessità di mantenere in capo agli Stati membri un certo grado di flessibilità nelle proprie scelte di politica economica e di bilancio e nel modo più trasparente possibile. Dopo che il Governo si è espresso, questa è e sarà la sede dove quelle politiche economiche e di bilancio verranno approvate e controllate. Il successo italiano in sede di *task force* ha determinato l'inclusione di parametri tipicamente italiani, perché questo vuol dire difendere il nostro specifico:

che ci consentono di affrontare ancora il peso della crisi finanziaria, ad esempio sul costo del debito pubblico, e devono consentirci di affrontare negli anni che sono davanti a noi tutti quei parametri e quei valori

Sono conclusioni importanti, quelle della *task force*, che attendiamo e che probabilmente porteranno, come dicevo prima, la stessa *task force* al tentativo di rivedere una parte del Trattato di Lisbona, proprio per rendere più cogente questa nuova impostazione di *governance*. Infatti, anche il meccanismo di sorveglianza

Van Rompuy - di bolla immobiliare o di modelli insostenibili per la bilancia dei pagamenti, ovvero di forti divergenze nella competitività. Tipologie di rischio trascurate nel primo decennio di vigenza dell'euro, quel primo Trattato di Maastricht che sta dietro a noi. conclusioni mitigano e hanno mitigato l'eccessiva rigidità con la quale era stata predisposta la proposta dalla Commissione: basti pensare, ad esempio, ai meccanismi più flessibili relativi alle misure di "allerta" e di "sanzione". Certamente restano da chiarire le modalità di calcolo e gli specifici criteri quantitativi e tecnici con i quali sarà ritmato il rientro, ma un'opportuna flessibilità rappresenta un'importante conquista e non solo per l'Italia. Essa ha evitato ed eviterà di fondare l'intero impianto di questa nuova *governance* su criteri numerici artificiosi, impossibili da rispettare, così da dover replicare per essa l'aggettivo di «stupido», con il quale, in più occasioni, autorevoli esponenti politici ed economici hanno bollato il Patto che avevamo sottoscritto È stato giusto, quindi, da parte dei Ministri dell'economia non affidare il percorso di rientro a rigidità e automatismi che avrebbero comportato inevitabilmente ritmi insostenibili, misure coercitive che avrebbero indotto manovre recessive che spingono inevitabilmente verso la deflazione. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi della Commissione bilancio

per il paziente lavoro svolto nell'elaborazione della proposta di risoluzione, ricordando che la *task force* ha risposto riportando in capo alla politica la centralità delle scelte, non lasciandola alle burocrazie e non esautorando la sovranità dei Paesi membri. Ecco perché davanti a noi c'è Maastricht 2, e la sfida che sapremo cogliere a cominciare da subito, dal pronunciarsi su questo atto che fornisce al Governo la necessaria copertura per continuare sulla strada che ha percorso fino ad ora e ha portato a soluzioni complessivamente positive per il nostro Paese, quella che fornisce all'Esecutivo il mandato più ampio a trattare in sede europea per rendere le nuove regole comunitarie più sostenibili e compatibili con la situazione economica e sociale del nostro Paese.

alcunché in merito alla procedura successiva, e quindi ai pareri che verranno dati sui singoli regolamenti dalle competenti Commissioni. Venendo al merito della questione, abbiamo due argomenti di fondo: da un lato, il tema delle nuove regole di *governance* e la credibilità che va recuperata a livello di regole; dall'altro, il rinnovato ruolo della politica sulla burocrazia. Diversi colleghi hanno toccato in particolare questi due temi.

del percorso che di fatto ci obbliga a una politica di rigore seria e anche di riforme e di sviluppo e, nello specifico, il tema di come ristabilire credibilità al meccanismo di *governance* (quindi regole chiare e sanzioni chiare). L'intervento della senatrice Leddi, in particolare, ha posto l'accento sulla situazione della Non ci fosse stata la situazione di crisi generale, al 99 per cento si sarebbe andati verso una ristrutturazione del debito, una situazione di uscita normale da una situazione di di stress del debito sovrano. Nel contesto dato, invece, si è dovuto agire in un certo modo. Questo comporta due ordini di rischio: il rischio di stress sui mercati finanziari se le regole non sono chiare e certe e il rischio di azzardo morale da parte dei singoli Governi (perché tanto si sa che qualcuno interviene in ultima istanza). È evidente che i nuovi meccanismi di *governance* che si stanno mettendo in atto difficoltosamente e in tempi rapidi vanno proprio nella direzione di evitare entrambi questi rischi: cosa non semplice, e lo sappiamo. Il senatore Morando ha evidenziato molto approfonditamente il tema del coinvolgimento corretto che deve esserci da parte dei singoli Parlamenti nazionali, e il dibattito di oggi, di oggi, onestamente e modestamente, ha riportato fortunatamente ad intera evidenza per tutti i colleghi l'importanza di questo tema che altrimenti rischia di passare sotto traccia, poiché i giornali - lo abbiamo ascoltato prima nell'intervento del collega Rutelli - si occupano di tutt'altro, quando nel resto d'Europa invece questo è il tema all'ordine del giorno, come anche il collega Legnini ha giustamente sottolineato. La seconda questione è relativa al ruolo dei singoli Parlamenti, della politica con la «P» maiuscola, contrapposto al ruolo della tecnocrazia e della burocrazia. Diversi colleghi hanno evidenziato anche questo tema, in particolare i senatori Lannutti, Giaretta e Mascitelli; quest'ultimo giustamente ricordava la titolarità della politica in scelte che necessariamente si riveleranno anche dolorose e non semplici.

da un lato, pone tutti nella consapevolezza dell'importanza del tema; dall'altro, pone anche il Governo - come dimostra la presenza e l'impegno del sottosegretario Casero, che ha da subito accettato anche la metodica di questo dibattito - nella giusta responsabilità di rapportarsi correttamente con il Parlamento su questo tema.

d'impegno affinché si riesca a rispettare i tempi europei, che spesso non sono coincidenti con le normali prassi parlamentari.

ma ancora più complicato è tenere sotto controllo l'evoluzione della spesa, per come ci viene prospettata dai documenti europei. Analizzando in retrospettiva cosa è successo negli ultimi dieci anni, sarà sicuramente molto difficile contenere l'evoluzione della spesa così fortemente come ci viene richiesto; ancora più difficile sarà rientrare dal debito. questo metterà tutti nella condizione di scegliere una volta per tutte le priorità. Posto un tetto di spesa serio e ineludibile,

oggi e ieri abbiamo dibattuto approfonditamente un'altra cosa, ossia la *governance* europea. Chiederei, quindi, al senatore Rutelli un'ulteriore riflessione in questi momenti, se possibile coodinandosi anche con con gli altri Gruppi, affinché non si sprechi un'occasione. Questo è il punto. Abbiamo dibattuto della *governance* e trovato una soluzione condivisibile e unitaria. Sarebbe uno spreco e un'occasione persa portare in votazione una mozione che è importante ma che però affronta altri argomenti, che non abbiamo oggettivamente dibattuto, quali

dal punto di vista sostanziale; sarebbe meglio aggiornarne la votazione ad un'altra sede, in modo che ci sia la possibilità di arrivare a un dibattito approfondito e quindi ad una votazione consapevole.

all'inizio un invito al ritiro, in quanto assorbita, con la richiesta, se gradita, di aderire, anche da parte

devo dire, è stato molto produttivo e utile sia per la posizione che il Governo dovrà portare al vertice europeo di oggi e domani, che per il futuro sviluppo del Paese. Queste decisioni che vengono prese in Europa in questi giorni nascono da un evolversi immediato e veloce di crisi finanziaria

pesante momento di crisi che è stato superato attraverso un'azione condivisa. Questa situazione nasceva dalla debolezza di uno dei Paesi europei, la Grecia, che aveva mostrato tutta una serie di inadempienze e di errori nella politica economica economica di gestione del Paese stesso, ma anche da una serie di debolezze insite nel processo di unificazione europea. Nel passato, si è pensato di arrivare a un'unificazione europea attraverso una serie di passaggi, che però spesso non hanno avuto una loro conseguenza logica, cioè un passaggio successivo. si è fatta l'unione doganale e poi si è capito che senza una moneta unica non poteva esistere un'unione doganale seria. In questi giorni si sta comprendendo che non è possibile mantenere una moneta unica senza una politica economica unitaria e una politica di bilancio convergente. Senza questi elementi non è possibile proseguire nel processo che tutti vogliamo di unificazione europea. I Governi europei, con tempi e metodi europei - quindi molto veloci, vista anche la gravità della crisi - stanno procedendo a passi forzati su un processo di unificazione delle politiche di bilancio. Riteniamo che ci debbano essere anche in seguito passi successivi che possano avvicinare i Paesi verso politiche di competitività e

possibile proseguire in questo processo, che deve essere spedito. Dicevo che con tempi e metodi europei è stata velocemente creata una commissione, che ha presentato un piano, e si è svolta una serie di incontri fra Governi per proseguire su questa tutto questo processo presenta dei limiti, che sono stati evidenziati nei vari interventi.

senza mischiare situazioni di debolezza o debiti dei vari Paesi, si possa perseguire una politica di infrastrutturazione europea attraverso l'emissione di titoli europei può essere uno degli obiettivi che si deve dare l'Europa nel momento in cui decide di avere una politica economica di sviluppo. Naturalmente, il dibattito è partito a livello europeo cercando di intervenire immediatamente su quello che è ritenuto da tutti come il principale elemento di debolezza finanziario dei singoli Paesi: l'eccessivo debito pubblico. Il dibattito in una prima fase era stato legato solamente agli obiettivi e ai tempi di rientro del debito pubblico,

non coerenti con uno sviluppo della finanza pubblica possano incidere pesantemente sullo sviluppo complessivo di una stabilità europea. Un altro obiettivo che dobbiamo porci è far sì che si consideri una molteplicità di fattori per le scelte di politica economica e non solo il fattore, che comunque è prioritario, della riduzione del debito. Tornando alla partita della riduzione del debito, che, ricordiamolo, è il principale obiettivo su cui l'Europa in questi giorni si sta interrogando e su cui sta decidendo (molto probabilmente prenderà decisioni che diventeranno cogenti per le nostre scelte future), si dovrà cercare di definire la percentuale di rientro e i tempi di rientro da una situazione attuale di eccesso di debito pubblico. Questa è un'altra delle partite che vengono giocate in questi giorni e che verranno giocate nei giorni successivi in Europa, sapendo però che il rientro del debito pubblico è un obiettivo imprescindibile sia per il nostro che per tutti i Governi europei. La funzione di questo dibattito che si è svolto in Aula e di questa proposta di risoluzione che verrà votata oggi è fondamentale, per una serie di ragioni. Innanzitutto, permette al nostro Paese di arrivare in Europa con una soluzione più forte. Spesso, troppo spesso, nel passato siamo arrivati divisi in Europa, e queste divisioni sono costate in termini di rapporti e di decisioni: sicuramente ci hanno danneggiato. In secondo luogo, anche in chiave interna, se questo Parlamento, se l'intero Paese, e anche i media - sono stati chiamati in causa perché hanno dato poco risalto a questo dibattito - capiscono che

di prendere una serie di decisioni che potranno essere produttive per il nostro sviluppo. Quindi, tutti i discorsi fatti in termini di competitività del Paese, di interventi infrastrutturali e di interventi su decisioni che sono

questo Paese deve proseguire, stimolare una politica di riforme che possa permetterci di competere nel modo migliore con gli altri Paesi, eliminando una serie di squilibri

Presidente, abbiamo esaminato questa mozione per una decisione che è stata presa sull'urgenza delle esigenze del calendario da parte della Conferenza dei Capigruppo. È chiaro che questa mozione tocca tematiche diverse da quelle su cui è stato messo principalmente l'accento oggi, cioè le questioni della crescita dell'economia, piuttosto che le esigenze della stabilità, che sono l'oggetto di una proposta di risoluzione che, lo preannuncio,

se infatti dovesse finire nella stessa condizione di incertezza nella quale si è trovata nelle precedenti settimane, meglio varrebbe concluderne l'esame oggi con una votazione.

ringrazio il presidente Rutelli per questa sua disponibilità a trattare in un'altra sede, in sede propria, la sua

la crisi economica e finanziaria internazionale ha messo a nudo la fragilità delle finanze pubbliche in diversi Paesi dell'Unione europea e dell'area dell'euro. Alcuni Paesi, come la Grecia, la scorsa estate hanno sfiorato il *default* facendo temere per la tenuta stessa della moneta unica. Sappiamo tutti che la crisi dei mercati finanziari internazionali è stata soltanto il fattore scatenante di questa situazione, perché le vere cause sono le criticità pregresse nelle finanze pubbliche di questi Paesi. Queste criticità risiedono non soltanto nella gestione finanziaria vera e propria, cioè nel modo in cui vengono impiegate le risorse pubbliche in quei Paesi, in poche parole come si usa la spesa pubblica e quanto si spende in rapporto al gettito fiscale. C'è anche un altro aspetto critico, che riguarda la trasparenza, la veridicità e l'affidabilità dei bilanci pubblici nei Paesi che aderiscono all'euro. Le regole del vecchio Patto di stabilità e crescita, che pure hanno consentito ai Paesi membri di convergere verso la moneta unica, alla lunga, si sono mostrate dunque non idonee a garantire la trasparenza dei conti pubblici e la definitiva stabilizzazione delle finanze pubbliche europee. Nemmeno esse sembravano in grado di governare il rientro dei deficit pubblici dopo che in molti Paesi questi ultimi sono cresciuti a causa della maggiore spesa pubblica erogata con i piani di sostegno alla finanza e all'economia reale colpite dalla crisi economica globale. Per questo, in sede europea si è reso necessario mettere mano al vecchio Patto di stabilità e crescita modificando le regole preesistenti e introducendone delle nuove. Il principio ispiratore dell'attuale riforma della *governance* europea, come nel precedente Trattato di Maastricht, continua ad essere quello secondo cui l'equilibrio e la solidità della finanza pubblica sono prerequisiti per la crescita economica. Principio, che in termini pratici, per i Paesi membri si traduce nella applicazione di una sola regola: il rigore finanziario. Ecco allora che, le nuove regole diventeranno presumibilmente più stringenti. Esse non riguarderanno più soltanto la gestione dei bilanci pubblici, ma sono destinate ad investire decisamente anche l'ambito più generale della politica economica. Le proposte di regolamento della Commissione, infatti, riguardano l'aspetto della prevenzione e della correzione sia degli squilibri dei conti pubblici sia degli squilibri macroeconomici. Insomma, siamo a un momento di svolta importante per la politica economica e finanziaria in Europa e di conseguenza in Italia. Con questa riforma della *governance* economica dell'Unione europea disegnata nelle proposte della Commissione si interviene in modo molto incisivo sulla discrezionalità dei Paesi membri in tema di politica di bilancio e di politica economica. Ciò risulta ancora più evidente se si pensa che, con l'introduzione del semestre europeo, i nostri documenti di bilancio dovranno, oltre che coordinarsi con lo scadenzario a livello dell'Unione europea, anche recepire le linee programmatiche dettate a livello europeo. Questa è una cosa di non poco conto, non solo perché ci costringerà a rivedere le scadenze della nostra sessione di bilancio appena riformata con la nuova legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009) per coordinarle meglio con quelle europee, ma anche perché dovremo ridisegnare anche tutte le scadenze relative ai dati statistici economici e finanziari rilasciati dalle istituzioni preposte, affinché essi siano disponibili per tempo e nella qualità necessaria a redigere documenti programmatici chiari, trasparenti e costruttivi. Ricordiamo che questo è un requisito essenziale per consentire al Parlamento di essere informato sulla situazione economica del Paese e di esprimersi sul merito in modo propositivo ed efficace. E allora vogliamo richiamare l'attenzione di questa Assemblea sulle conseguenze per un Paese come l'Italia per un Paese come l'Italia derivanti da una impostazione, quale quella della Commissione europea, ispirata al solo principio del rigore finanziario. Voglio richiamare in proposito quanto detto dal collega Baldassarri nella seduta di ieri, circa la necessità che l'Europa si preoccupi non solo del rigore finanziario, ma anche dello sviluppo e della crescita dell'economia e quindi delle prospettive dell'occupazione. Perché se è vero che l'equilibrio e la stabilità delle finanze pubbliche sono una condizione importante e necessaria per garantire una crescita solida dell'economia, è anche vero che pensare di conseguire l'equilibrio e la stabilità della finanza pubblica

In questo senso - secondo noi - l'Italia, con il suo Ministro dell'economia, deve lavorare e far sentire la propria voce presso le istituzioni europee. Ripetiamo: non la sola gamba del puro rigore, ma entrambe le gambe del rigore e della crescita. Da questo punto di vista, per quanto riguarda sia la perdita di discrezionalità che si profila all'orizzonte, che per l'eventualità che le regole del nuovo Patto europeo di stabilità e crescita vengano costruite su semplici automatismi aritmetici, basati sul solo deficit complessivo e sul livello del debito, l'Italia rischia di essere penalizzata. È importante che in sede di discussione delle nuove regole si arrivi a introdurre meccanismi più flessibili, che tengano conto ragionevolmente delle condizioni più generali dell'economia italiana. Ecco allora che è importante che si tenga adeguatamente conto di altri parametri, quali lo stato di salute del settore privato e del risparmio complessivo nazionale. Dunque, in conclusione, a fianco di un convinto voto favorevole, il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia pone al Governo le prescrizioni politiche di cui sopra e chiede che ci si faccia con chiarezza sentire in ambito europeo,

la convergenza e il nostro voto favorevole sulla proposta di risoluzione n. 3, che è stata il risultato di un impegnativo e intenso lavoro compiuto compiuto da tutti i componenti della Commissione bilancio, sotto la guida del presidente Azzollini, al quale va tutto il nostro ringraziamento. È una proposta di risoluzione che si muove su alcune direttrici che abbiamo sempre considerato estremamente importanti, tra della trasparenza dei dati, delle informazioni e delle valutazioni. Ora, questa trasparenza non viene più chiesta soltanto dall'opposizione,

che l'importante Piano nazionale di riforma sia discusso in questo ramo del Parlamento nei prossimi giorni. La proposta direzione della sovranità del Paese. In questo momento il Parlamento è unito per cercare di riaffermare la sovranità del ruolo del Paese del Paese nella scelta delle politiche nazionali. In questo senso ci siamo mossi ormai già da tempo. Ricordo che una proposta di risoluzione con analoghi contenuti

Detto questo, signor Presidente, mi consenta anche di chiarire alcune considerazioni, cioè chiarire lo spirito con il quale il Gruppo dell'Italia dei Valori si appresta a votare questa proposta di risoluzione unitaria.

l'alibi per cui tutto quello che si fa nel nostro Paese ci è chiesto dall'Europa. L'Europa ci chiede la stabilizzazione dei conti pubblici, ci chiede il controllo e la sorveglianza dei conti pubblici; ma

Così come l'Europa non ci ha mai chiesto, a fronte dell'operazione (da noi definita senza alcuna polemica vergognosa) dello scudo fiscale tassato al 5 per cento, che l'aliquota di tale tassazione dovesse essere così tanto inferiore rispetto a quella di altri Paesi europei, compresa la Germania.

cui in tempi di crisi non sarebbe consentita la crescita. Anche questo aspetto deve essere finalmente chiarito: gli Stati membri hanno sottoscritto l'Agenda 2020, che sarà il prossimo campo di sfida per le scelte future, nella quale la stabilizzazione dei conti pubblici va di pari passo in termini di rafforzamento e di sostegno con le politiche della crescita. E forse, tutto sommato, l'Agenda di Lisbona, ormai arrivata alla sua scadenza, è fallita per i suoi contenuti in non è riuscita a creare quegli incentivi per poter favorire e sostenere la politica della crescita. Non è più possibile, quindi, usare questo alibi,

Non è dell'anno scorso, ma soltanto di pochi giorni fa, una graduatoria stilata da un organismo terzo, il *World economic forum* che pone il nostro Paese in termini di competitività al 48º posto, dopo la Tunisia, la Lituania e l'Estonia. Su questi aspetti dobbiamo riflettere e affrontare come Parlamento le scelte future che ci attendono. Lo Lo diciamo oggi come lo abbiamo detto in questi due anni: in termini di crescita economica e di competitività del nostro Paese, le misure che questo Governo ha avuto la capacità di mettere in atto sono state poche, poche, inadeguate e insufficienti. Rispetto alla crisi delle imprese e alla necessità che le piccole e medie imprese avessero un sostegno alla loro crescita e al loro sviluppo, abbiamo assistito

zero", presentata dal Ministro dell'economia, anche in sede di audizione, come elemento di grande strategia politica nazionale, addirittura da prospettare come esempio all'Europa. piuttosto che le piccole e medie imprese del nostro Paese, che vivono un problema di "mortalità" particolarmente accentuato, abbiano bisogno non non tanto di semplificazione, ma piuttosto di supporto alla crescita, cosa che non è mai stata fatta in questi due anni di politica.

di questo dato, però, cerchiamo di considerarne anche un altro, estremamente utile per comprendere la disuguaglianza sociale in cui vive il nostro Paese:

Lo diciamo al ministro dell'economia Tremonti, oggi impegnato al vertice...

erano i numeri che andavano dietro la politica, ora è la politica che deve andare dietro i numeri. Vorremmo che la politica andasse dietro i bisogni e le attese della gente.

senza che il Parlamento e forse - mi permetto di dire, come ho già fatto in Commissione - neanche il Consiglio dei Ministri siano stati investiti della discussione preliminare necessaria ad affrontare le decisioni

il piano delle riforme che la nuova *governance* gli impone di presentare il prossimo 10 novembre, cioè Saremmo arrivati a quell'appuntamento dando tutto per scontato; invece è bene che nella risoluzione sia scritto che noi sul merito facciamo un dibattito. Questo è uno dei punti

sul versante politico; a tale riguardo mi dispiace che, invece, i contenuti della risoluzione approvata all'unanimità in Commissione esteri sotto la guida del presidente Dini, che da questo punto di vista erano un po' più pregnanti, un po' più aggressivi, siano stati in qualche modo ridotti nella loro importanza nella proposta di risoluzione finale che è in votazione. Lo sottolineo perché in realtà, e su questo aspetto vorrei soffermarmi qualche minuto, la questione non è tecnica: è tutta politica. La grande paura che ha colpito i Paesi dell'Unione, a partire da quello più ricco, durante l'ultima crisi che abbiamo attraversato (quando veniva persino messa in dubbio la possibilità che la moneta unica reggesse l'impatto con la speculazione che si stava scatenando in quei giorni, in quelle ore), quella grande paura ha fatto fare un balzo alla politica dell'Unione europea, determinando quel fenomeno che ricordava così efficacemente il collega Tonini che portava gli Stati fino a prima della crisi a rinchiudersi nelle proprie frontiere e ad inseguire l'Europa minima indispensabile a rilanciare per forza il ruolo dell'Europa, improvvisamente, senza avere però avvertito le loro opinioni pubbliche che questo processo si stava determinando. In realtà vi è un paradosso:

stare tranquilli, perché i numeri non sono rigidi, c'è flessibilità. Dobbiamo smetterla di discutere di cose così importanti dicendo che dobbiamo approvarle perché ce le impone l'Europa. Dovremmo provare a rovesciare decidiamo noi, insieme all'Europa, cosa è bene fare per l'Italia e per l'Europa. Non ritroviamoci come in occasione dell'ultimo decreto-legge che ha tagliato

d'ora in avanti questo atteggiamento, perché diversamente ci sarà chi deciderà per noi, e deciderà per noi il Paese più forte. forte. Non vorrei che fosse sfuggito il contenuto politico del vertice che si è svolto tra la Merkel e Sarkozy soltanto pochi giorni fa, alla vigilia del Consiglio che si svolge oggi e domani, nel quale i due Paesi - che come ricorderete hanno avuto qualche momento di freddezza nel passato più recente - hanno ritrovato improvvisamente una spinta unitaria, all'insegna "ci mettiamo noi a trainare e a decidere che cosa è meglio per l'Europa, gli altri ci devono stare per forza". Noi dobbiamo avere la consapevolezza che questa è la partita che si sta giocando nella dimensione politica europea, europea, decidendo cosa dobbiamo fare per essere all'altezza della dignità di un Paese fondatore che partecipa alle decisioni rappresentando uno dei grandi Paesi, sicuramente con alcune difficoltà, ma avendo la forza politica

agli *eurobond*. Badate che, a seguito della crisi della Grecia (che si è risolta con un pacchetto di risorse che ogni Stato membro ha messo a disposizione per fare un prestito alla Grecia), nelle nuove proposte è prevista l'istituzione di un fondo, ancora non del tutto definito, al quale affluiranno risorse dei Paesi membri, ma anche di privati: un fondo al quale si vuole dare una sorta di cittadinanza un po' strana. Ma per quale ragione non dobbiamo chiedere - come ha detto il ministro Tremonti in più occasioni - che venga ripresa pienamente la proposta del presidente Delors *(Applausi dal Gruppo PD)* e venga rilanciato il sistema degli *eurobond*, degli *eurobond*, avanzando l'idea di un prestito che consenta di intervenire nelle infrastrutture, ma anche verso i Paesi che dovessero trovarsi in difficoltà, così come è capitato alla Grecia? Ecco, questi sono i punti, su cui abbiamo avviato

(ma l'aspetto politico prevale sul resto) è che, dopo avere votato qui in Senato all'unanimità nel corso dell'esame della legge di contabilità l'istituzione dell'autorità indipendente sul *budget*, mi pare si stia facendo un passo indietro Siamo diventati timidi? Come mai il Senato ritorna su una decisione unanime assunta non molto tempo fa? Attenzione che qui c'è un rischio:

ancora una volta - sulla nostra testa e ci ritroveremo nella condizione di dover dire «lo dobbiamo fare perché ce lo chiede l'Europa». In conclusione, dichiaro il nostro voto favorevole alla risoluzione unitaria proposta,

perché l'Italia - qui siamo nel Parlamento italiano - partecipi a pieno titolo, e non solo formalmente, alle decisioni per disegnare il futuro dell'Europa, che sarà anche il futuro dell'Italia. *(Applausi

contribuire a dare una soluzione al tema della *governance* europea, alla necessità di avere non solo la moneta unica ma anche, per forza, il governo unico dell'economia. Signora Presidente, preannuncio il voto favorevole del Popolo della Libertà.

sulla condanna a morte dell'ex vice primo ministro iracheno Tareq Aziz. Ha facoltà di

una pesantissima sensazione.

È una pesantissima sensazione di ritorsione, vendetta e motivazione politica ad accompagnare la decisione di condanna all'impiccagione per Tareq Aziz e altri alti funzionari del passato regime iracheno. Dico questo senza nulla togliere alle ragioni di principio che hanno accompagnato anni di lotta politica (radicale e non solo) dei Governi e dei Parlamenti del nostro Paese, fino ad arrivare alla risoluzione delle Nazioni Unite per la moratoria della pena di morte, decisa nel 2007. Queste ragioni di principio e di legalità, volte ad evitare qualunque confusione tra giustizia e vendetta, rimangono

venuta immediatamente e che ci ha consentito di presentare d'urgenza una mozione, corredata dalle firme di numerosissimi colleghi di tutti gli schieramenti politici in questa Aula del Senato e alla Camera dei deputati. Ma voi mi consentirete anche di aggiungere che, oltre a tale questione di principio, accompagna questa dichiarazione di esecuzione la pesante sensazione di motivazione politica e di ritorsione. Ognuno di noi può avere le valutazioni più diverse rispetto al ruolo, le responsabilità di Tareq Aziz ed altri. Ma rimane il fatto con cui si è svolto il processo, nella opacità più totale, anzi nell'impossibilità persino degli avvocati difensori di seguire il processo, processo, ci portano davvero ad essere sempre più convinti che alle ragioni di principio si aggiungono, per quanto ci riguarda, anche

Penso che tutti dovrebbero, con grande prudenza e senso di responsabilità, verificare quei documenti e le informazioni che vi si trovano.

mi sembra che ogni giorno di più scopriamo lati oscuri e terribili, sia in ordine all'entrata in guerra e alla dichiarazione di guerra decisa nel marzo 2003, agli episodi terribili di quella guerra. E sempre di più, nel mondo intero, si alzano le voci che chiedono la verità su tutto quel periodo, perché la forza della verità è la forza delle democrazie, cioè di quei sistemi che sanno correggere i propri errori quando li riscontrano, che sanno anche chiedere le dimissioni, per esempio, dei più alti esponenti politici, quando si scopra che si sono macchiati di reati. Questa è la forza della democrazia, di quel sistema che sa fare della verità un momento di correzione dei suoi errori e dei momenti più oscuri. Tareq Aziz è indubbiamente quasi l'ultimo testimone, possibilmente scomodo, di tutta quella vicenda, di tutti quei retroscena che ancora non sappiamo. Forse anche per questo la sua condanna improvvisa: i colleghi sanno ad esempio che proprio due settimane Tareq Aziz era stato prosciolto dalle accuse mossegli in un altro processo che aveva in corso. La sensazione - per quanto mi riguarda, la convinzione - è che la sua messa a morte sia anche un modo di eliminare l'ultimo testimone forse scomodo, ma che certamente certamente sa molte cose che sarebbe bene sapessimo tutti, soprattutto noi, che ci vantiamo di vivere in Paesi democratici. Noi radicali continuiamo ad essere convinti ed abbiamo continuato a documentare che era possibile sostenere l'azione diplomatica dei Paesi del Golfo per l'esilio forzato di Saddam Hussein abbiamo continuato a darne conto e prova, fino alla dichiarazione del Bahrein, che si diceva disponibile ad ospitare Saddam Hussein. Il Parlamento italiano, l'unico Parlamento al mondo, chiese con grande forza che questa ipotesi venisse perseguita, perché questo avrebbe consentito che un dittatore sanguinario uscisse dal proprio Paese per consentirne un'evoluzione diversa, senza un atto di guerra che molti hanno giudicato illegale e che comunque ancora oggi presenta lati di motivazione che non sono stati chiariti. Forse anche nel nostro Paese e in questo Parlamento sarebbe utile una Commissione d'inchiesta. Ripeto, conoscere la verità, ammettere ciò che non si è voluto o potuto fare, è uno dei deterrenti più straordinari per non ripetere gli stessi errori. Noi radicali siamo persone che credono nella non violenza, e non nel pacifismo, che fa una certa differenza (su cui oggi non mi dilungherò): è un'altra cosa. Non abbiamo sfilato con milioni di persone contro la guerra: abbiamo lottato per altro, affinché l'iniziativa diplomatica dell'esilio forzato trovasse sufficiente supporto diplomatico contro le decisioni prese tempo prima da Bush, da Blair, da altri e sostenute anche dal nostro Governo dell'epoca. Questa era la strada che avremmo dovuto percorrere. Oggi continuiamo a chiedere la verità. La forza del *satyagraha*, della verità, della non violenza ha portato e porta Marco Pannella ad essere al secondo giorno di sciopero della sete. So che c'è chi ne sorride e chi apertamente deride; pregherei invece tutti di fare attenzione al merito delle cose che vengono chieste oltre che allo strumento con cui vengono chieste. Quello che chiediamo è una grande azione diplomatica affinché nessuno tocchi, non solo Caino, ma neanche Tareq Aziz e gli altri, e sottolineo «gli altri». Oggi, nel nuovo regime iracheno, così fragile e debole, che non riesce neanche dopo sette mesi a costituire un Governo,

come lo abbiamo chiesto agli amici americani per Teresa Lewis, inascoltati, chiediamo una grande azione diplomatica perché ne sia evitata la messa a morte e questo contribuisca ad un'estensione della moratoria. Ricordo che, subito dopo la caduta del regime, l'Iraq decise la moratoria sulla pena di morte; questa moratoria è stata rinnegata e ritirata solo poco tempo fa. fa. Credo che la forza di un Paese democratico, del suo Governo e delle sue istituzioni sia anche quella di riuscire ad andare, quando necessario, controcorrente controcorrente rispetto agli alleati. Credo, infatti, che la forza delle convinzioni sia anche la forza nobile di una politica, in particolare, e non solo, a livello internazionale. Per tutti questi motivi, e sapendo che altri colleghi hanno magari altre motivazioni *ad adiuvandum*, con grande convinzione, signori del Governo, vi chiediamo di mettere in moto tutto quanto è possibile affinché questo nuovo obbrobrioso assassino, insieme con tutti gli altri,

Spero che voteremo la mozione tutti insieme e che questa forza di unità istituzionale dia anche al Governo la forza di interloquire rispetto a grandi alleati,

Signor Presidente, credo che la Lega Nord possa a buon diritto considerarsi al di sopra e al di fuori di ogni sospetto buonismo o equivoca indulgenza nei confronti dei nemici dell'Occidente; nondimeno, quel senso di giustizia e umanità che non può fare difetto in chi guarda ai valori più radicati nella nostra gente ci motiva a unirci senza indugio a quanti,

ha già suscitato, tra le altre, le prese di posizione dell'Unione europea, della Presidenza della Repubblica italiana e del Vaticano, ed è doveroso che la questione venga affrontata anche in questo consesso. Si tratta manifestamente di un caso politico di grande portata: lo attesta il ruolo ricoperto da Tareq Aziz nel contesto dell'Iraq di Saddam Hussein e lo evidenzia la mobilitazione promossa intorno al nome di questo personaggio dai fautori dell'abolizione della pena di morte. caso politico, come dicevo: certamente non avrebbe suscitato le stesse premure il destino di uno dei sette sconosciuti compresi nella media quotidiana delle esecuzioni capitali nel mondo. In gioco, invece, c'è la vita di un uomo che nel corso della sua carriera è stato ai vertici di una Nazione incontrando governanti di molti Paesi, e persino il Papa. Tanto la forza quanto la debolezza di questa causa risiedono precisamente nella trasposizione del dramma personale a un fatto di bandiera, criterio espresso nell'editoriale del più importante quotidiano nazionale, dove si afferma che un comandamento universale iscritto nell'identità forgiata dai Lumi impone di rispettare i diritti umani anche di chi ne ha fatto scempio nel modo più grave. Dunque, a Tareq Aziz, benché correo dei peggiori crimini e meritevole delle sanzioni più severe, dovrà essere risparmiata la pena di morte perché retaggio di secoli bui. A parte il fatto che la Nazione culla dell'illuminismo tenne bene oliata la ghigliottina fino al 1981, ritengo discutibile, oltre che controproducente ai fini della sua salvezza, accettare acriticamente la criminalizzazione dell'ex Vice *Premier* iracheno. Diritti umani non significa solo ergastolo invece della forca: vuol dire anche il diritto ad un equo processo, e questo, per Tareq Aziz, non vi è stato. Il suo avvocato italiano si è lamentato di non aver neppure potuto formulare una domanda ai testimoni. Aziz è stato condannato a morte perché incolpato della persecuzione compiuta dal regime contro il partito sciita, ma lo stesso difensore ha specificato che il suo assistito aveva partecipato non più di due volte in ventisei anni alle riunioni del consiglio rivoluzionario, l'organismo responsabile della politica interna irachena. Pare che Tareq Aziz, infatti, si sia pressoché esclusivamente occupato dei rapporti con i Paesi stranieri. Varrebbe la pena di spendere due parole su questa figura di politico, direi anomala nel panorama degli Stati islamici. Questo uomo di 75 anni, oggi in precarie condizioni di salute e reduce da sette anni di detenzione, decisamente non rispecchia lo stereotipo dell'integralista fanatico, fiancheggiatore del terrorismo internazionale. Cristiano, di rito caldeo, Chiesa locale in unione con il Papa, l'ex Vice *Premier* iracheno si dimostra un sincero estimatore della cultura europea. Intrattiene intensi rapporti diplomatici con diversi Paesi occidentali, frequenta volentieri le città del Vecchio Continente. Lo ricordiamo in ginocchio davanti alla tomba di san Francesco, ad Assisi, nel febbraio 2003; un mese prima dell'attacco all'Iraq, viene ricevuto in Vaticano da Giovanni Paolo II. La sua posizione influente ha contribuito a garantire alla minoranza cristiana irachena una situazione di prosperità e serenità del tutto invidiabile rispetto alla gran parte dei Paesi islamici. Evidentemente, fu uomo di potere, di sicuro al corrente dei rapporti intercorsi tra il regime di Saddam e i Governi occidentali. Pare, dunque, pienamente fondata l'osservazione formulata nella mozione radicale che l'impiccagione di questo testimone eccellente e, direi, scomodo impedirà la ricostruzione della verità storica sulle responsabilità interne ed esterne al regime di Baghdad. Condivisibile è dunque, oltre che auspicabile, la proposta di sollecitare un intervento del nostro Governo presso le autorità irachene allo scopo di fermare la mano del boia. Oltre a motivazioni ideologiche e alle opportunità relative all'inammissibilità della pena capitale, sarebbe conveniente che la richiesta italiana prendesse in considerazione il diritto dell'imputato Tareq Aziz

ci dia la facoltà di pretendere che il nuovo regime si discosti dagli errori e abusi del passato. Qualora risultassero chiaramente e pervicacemente disattese le condizioni minime di garanzia dell'imputato, più che alle istituzioni irachene sarebbe opportuno rivolgersi all'autorità americana, che ha in carico il detenuto, affinché Tareq Aziz non venga consegnato a una vendetta che di giustizia avrebbe solo il nome.

a parlare dei Caini di tutto il mondo, conosciuti o sconosciuti e, soprattutto, dei Caini che fanno parte dei peggiori regimi che hanno caratterizzato la seconda metà del secolo scorso. Mi riferisco ai regimi che hanno violato sistematicamente non solo i diritti umani, ma anche il diritto umanitario internazionale. Nel 2006, alla vigilia dell'esecuzione di Saddam Hussein, Marco Pannella entrò in sciopero della fame e sete per evitare che venisse ucciso uno dei peggiori dittatori di questi ultimi anni. Quell'iniziativa non riuscì a salvare la vita a Saddam Hussein, ma lanciò in maniera molto decisa la campagna che portò all'adozione della risoluzione del 2007 sulla moratoria universale della pena di morte. Nel luglio 2008, come l'altro ieri, ancora una volta la nonviolenza di Marco Pannella ha portato il Parlamento italiano (nel luglio 2008 con una lettera-appello firmata da tutti i presenti in Commissione affari esteri, oggi con questa mozione condivisa da quasi tutti i Gruppi, tranne la Lega) ad occuparsi di un Caino, e di altri due Caini non si parla soltanto di Tareq Aziz, come ricordava la senatrice Bonino in illustrazione del documento, ma anche di Saadun Shaker, ex ministro dell'interno, e dell'ex segretario personale di Saddam Hussein, Abdel Hamid Hamud - che sono stati condannati all'impiccagione.

veramente drammatico è riuscire a formulare un'espressione come quella della faccia presentabile di un regime perché forse, proprio grazie a questa faccia presentabile, si riesce a non affrontare nel merito ciò che quel regime ha ha fatto nei confronti dei suoi cittadini, di qualsiasi etnia o affiliazione religiosa essi fossero. Ho sentito parlare di nemici dell'Occidente. Non so chi siano tali nemici, ma sicuramente ve ne è uno che sta minando al nostro interno anche le democrazie liberali, ed è quello di non rispettare la legge, di non rispettare la legge, i patti e gli obblighi internazionali. La giurisprudenza internazionale negli ultimi anni ha considerato la pena di morte una violazione dei diritti umani e lo ha fatto attraverso una serie di decisioni prese dal Consiglio di sicurezza stesso quando ha creato i tribunali *ad hoc*; la comunità internazionale, proprio a Roma, nel 1998 ha adottato lo statuto della Corte penale internazionale, che non prevede la pena di morte per crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di guerra. Tutto ciò che deriva dall'intervento internazionale deve mantenere gli standard più alti di giustizia internazionale sia in termini di giusto processo e di accesso alla difesa, ma anche di comminazione delle pene, e la pena di morte non viene morte non viene riconosciuta da nessuno di questi documenti internazionali. Ci troviamo alla possibile vigilia di un'esecuzione di un testimone fondamentale non soltanto per le nefandezze del regime di Saddam Hussein, ma anche per come si è arrivati alla guerra. Il 14 febbraio 2003 Tareq Aziz era in Italia ad offrire il suo aiuto per cercare una soluzione per la crisi presunta relativa alla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. anno, marzo Camera e Senato, unici luoghi dove si fanno le leggi nel mondo, adottavano una risoluzione che dava mandato al Governo italiano di adoperarsi alle Nazioni Unite per scongiurare l'intervento militare, favorendo la possibilità di mandare Saddam Hussein in esilio. Il 22 febbraio in una riunione, dove erano presenti telefonicamente Blair e Berlusconi, e fisicamente Aznar e il presidente Bush, si discuteva della possibilità reale di poter mandare Saddam Hussein e i suoi in esilio in un Paese terzo, e vi erano state anche offerte di ospitare Saddam Hussein stesso. Alla riunione del 1° marzo della Lega araba a Sharm el Sheik tale proposta non fu inclusa all'interno della risoluzione finale perché Gheddafi e i reali sauditi iniziarono una serie di offese in riunione pubblica, che fecero proseguire la riunione in sede segreta affinché non si sapesse di una non concordanza su certi temi all'interno della famiglia araba. Noi oggi chiediamo al Governo di farsi portatore della richiesta del Parlamento - ricordo che ieri lo ha fatto la Camera dei deputati - relativamente alla sospensione della pena di morte per i tre condannati e per fare applicare una moratoria in Iraq. Quel che poi però successivamente dovrà essere portato all'attenzione del Senato è la richiesta di una Commissione d'inchiesta su come si è arrivati a far partecipare l'Italia - seppure in maniera anomala

la mozione sottoscritta da moltissimi colleghi di quasi tutti i Gruppi qui rappresentati è stata bene illustrata poco fa. Ci sono due aspetti

questo martoriato Paese si era in un primo momento riconosciuto nei principi della moratoria, che avevano ispirato la risoluzione del 2007, sembra invece orientato a distaccarsene nel modo più drammatico. Da questo punto di vista, stamattina la stampa internazionale, («Le Monde», ma anche la stampa anglosassone) insiste sull'aspetto che la presidente Bonino ha chiamato di ritorsione, di vendetta e di rappresaglia. però anche adombrato l'aspetto di eliminazione di un testimone scomodo di tante vicende, non solo di quella richiamata dal collega Perduca, per la quale è stato ricordato Marco Pannella, al quale ognuno di noi nella sua storia politica e personale ha guardato e guarda talvolta con dissenso politico,

sgradevole e, sotto certi aspetti, difficilissima, a livello di diplomazia tra i Governi. Del resto, è inutile negare che il giudice che ha pronunciato la sentenza di morte era, settimane addietro, un candidato non eletto alle elezioni del *premier* Maliki. un uomo di Governo attento ed esperto come Vincenzo Scotti potrà corredare l'iniziativa italiana anche di quei canali non

all'amico - se così posso dire - presidente Schifani, che oggi ha prerogative molto importanti, abbiamo conosciuto il presidente Talabani,

Quello che ci guida, visto che si è parlato di rivoluzione francese, è un esempio che viene dalla rivoluzione americana: altro che le qualunquistiche battute, pubblicate ieri su «la Repubblica», di Adriano Sofri. Un eroe della rivoluzione francese ed americana, il marchese di Condorcet,

nell'iniziativa radicale e nell'iniziativa italiana del 2007, che richiamiamo con forza all'attenzione del Governo, insieme ai colleghi dei vari Gruppi politici. *(Applausi dal

ringrazio lei e gli altri senatori per aver voluto presentare con grande tempestività la mozione relativa alla condanna a morte dell'ex vice *premier* e ministro degli affari esteri Tareq Aziz. Come sapete, un analogo testo è stato già approvato ieri alla Camera dei deputati. Anche qui, in Senato, la mozione che stiamo discutendo ha ottenuto un appoggio trasversale, il Governo intende esprimere un parere pienamente favorevole, perché è mosso dallo stesso spirito e dalla stessa determinazione che animano il Parlamento e la società civile italiana nel condurre battaglie di civiltà. Anche di fronte a questa immediata mobilitazione del nostro Parlamento sul caso dell'ex Ministro degli esteri iracheno, permettetemi di rinnovare - l'ho fatto ieri alla Camera dei deputati - all'amico Marco Pannella, che questa mattina è stato audito dalla Commissione esteri della Camera, l'appello di un amico a mettere fine allo sciopero della fame e della sete. Il 26 ottobre, l'annuncio della sentenza di condanna a morte di Tareq Aziz è stato dato dall'Alto tribunale iracheno nell'ambito del processo per le esecuzioni e le violenze ai danni di membri di partiti religiosi perpetrate durante gli anni del regime di Saddam Hussein. Con lui sono stati condannati anche l'ex capo dei servizi, Saadun Shaker, ed il segretario personale di Saddam, Abdel Hamud. La sentenza può essere appellata entro un mese. Trattandosi di condanna alla pena di morte, l'intervento di un'istanza superiore avrà comunque luogo automaticamente. La Corte di primo grado che l'ha pronunciata è formata da cinque giudici,

potrebbe quindi intervenire non prima di quattro o cinque mesi. Secondo la legislazione che disciplina l'Alto tribunale (Corte speciale istituita nel 2005 per i crimini di genocidio e contro l'umanità commessi in Iraq negli anni del regime), non è ammessa la grazia da parte del Presidente della Repubblica né occorre, come invece nelle condanne a morte per delitti comuni disciplinate dal codice penale ordinario, la sua firma sull'atto di esecuzione. La questione verrà quindi esclusivamente trattata, almeno sotto il profilo legale, in ambito giudiziario, senza il coinvolgimento dell'Esecutivo o di altra figura politica. Tutto si baserà conseguentemente sulla decisione del tribunale di appello, la cui ampia composizione potrà peraltro risentire di diversi orientamenti e sensibilità. Una legge del nuovo Parlamento, peraltro inattivo in ragione dello stallo politico in cui si trova il Paese, che doti il Presidente della Repubblica di un potere di grazia anche per i crimini in oggetto appare al momento più che improbabile. Sempre sul fronte politico, non va dimenticato che la condanna interviene in un momento delicato delle trattative per la formazione del nuovo Governo e rischia di non facilitare la riconciliazione nazionale e il consenso tra le forze politiche impegnate in un difficile negoziato che si protrae dal marzo scorso. Il presidente della Repubblica Napolitano ed il ministro Frattini, in visita ufficiale a Pechino, non hanno esitato ad associarsi alla presa di posizione da parte dell'Alto rappresentante UE, Ashton, la quale, a nome dell'Unione europea, ha fermamente condannato la sentenza capitale comminata a Tareq Aziz. L'alto rappresentante Ashton ha, infatti, annunciato l'intenzione di chiedere alle autorità di Baghdad di bloccare l'esecuzione, dal momento che la pena di morte "non è accettabile" per l'Europa. Come detto, si tratta di una posizione condivisa, a nome del Governo, dal ministro Frattini, alle cui dichiarazioni hanno fatto eco, tra gli altri, i miei colleghi Craxi e Mantica, che hanno sottolineato che la decisione del tribunale iracheno non va certo in favore della costruzione di un nuovo Iraq democratico ed è "assolutamente inutile". Un coro di no all'esecuzione è peraltro giunto anche dal Parlamento europeo. Parallelamente, il nostro ambasciatore a Baghdad è immediatamente intervenuto presso le autorità irachene e ha incontrato, subito dopo l'annuncio della condanna di Tareq Aziz, il Ministro dei diritti umani e il Vice Ministro della giustizia. Successivamente ha avuto un colloquio con il primo ministro Maliki, sottolineandogli la grande attenzione e la riprovazione con cui la questione è seguita in Italia e nel resto d'Europa, nell'opinione pubblica e parlamentare e anche ai più alti livelli istituzionali. L'ambasciatore ha ribadito la nostra posizione in materia di pena di morte e, nell'esprimere rispetto per l'ordinamento giudiziario iracheno e per le regole costituzionali e legislative che lo disciplinano, ha fatto stato dell'auspicio unanimemente diffuso in Italia, espresso dal Presidente della Repubblica e dal ministro Frattini, che l'esecuzione non abbia luogo e che la sentenza pronunciata in primo grado sia rivista, considerata anche l'età avanzata del condannato. Maliki ha ribadito la totale indipendenza della magistratura e ha affermato che non avrebbe certo obiettato ad una revisione della sentenza in appello. Il nostro rappresentante a Baghdad ha in programma di svolgere ulteriori sensibilizzazioni con altri esponenti iracheni, in particolare con il presidente della Repubblica Jalal Talabani. Talabani. A fronte del carattere esclusivamente giudiziario del procedimento, che deve peraltro ancora giungere a conclusione, l'azione del Governo italiano sarà volta a ricordare con forza alle istituzioni irachene che gli organi della magistratura coinvolti possono applicare la moratoria universale della pena di morte, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel dicembre 2007. Questo concilierebbe il necessario rispetto per la procedura tutta giurisdizionale, prevista da una legge applicabile nello Stato straniero, con l'aspettativa che il giudizio d'appello faccia proprie considerazioni, pure giuridiche, in cui si è andata traducendo la sensibilità ormai prevalente nella comunità internazionale. Questa azione si pone peraltro in linea con la politica estera italiana dei diritti umani, nell'ambito della quale l'abolizione della pena di morte nel mondo rappresenta una delle principali priorità. L'Italia, insieme ai partner dell'Unione europea e ad una vasta alleanza transregionale di Paesi, si è fatta promotrice, infatti, della già ricordata risoluzione sulla moratoria per la pena di morte del 2007, con 104 voti a favore, e, nel 2008, con 106 voti a favore. Come riconosce anche un recente rapporto sull'argomento del Segretario generale della Nazioni Unite, esiste una tendenza internazionale verso l'abolizione della pena capitale. Una tendenza che va ulteriormente consolidata, ed è quanto intendiamo fare con la risoluzione sulla moratoria della pena di morte che, insieme con i Paesi appartenenti a tutte le aree geografiche del mondo, stiamo discutendo anche quest'anno a New York, che verrà presentata nei prossimi giorni alla Terza Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e successivamente in plenaria. Stiamo negoziando per Stiamo negoziando per introdurre nella risoluzione di quest'anno alcuni aspetti che riteniamo rilevanti per ridurre l'applicazione della pena capitale nei Paesi che ancora la praticano. In particolare, abbiamo chiesto di inserire nel testo un espresso appello agli Stati a rendere pubblici i dati sulle condanne a morte e sulle esecuzioni, dal momento che proprio la mancanza di informazione dell'opinione pubblica sui "fatti"

avvicinandoci sempre più al traguardo ultimo dell'abolizione universale. L'impegno del nostro Paese a favore dell'abolizione della pena capitale si realizza anche attraverso un costante monitoraggio accompagnato da prese di posizione in relazione a casi individuali di condanne a morte. Con particolare riferimento all'Iraq, l'Italia ha recentemente raccomandato alle autorità di Baghdad, nel corso dell'esame periodico universale del Paese da parte dei Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (svoltosi a Ginevra nel marzo 2010), di reintrodurre una moratoria delle esecuzioni in vista della completa abolizione della pena di morte. La comunanza di intenti e la stretta collaborazione tra Governo, Parlamento e società civile italiana hanno sinora permesso - e continueranno a permettere, anche relativamente al caso di Tareq Aziz - all'Italia di portare avanti con successo questa battaglia, con un ruolo ed un impegno che le vengono universalmente riconosciuti. L'impegno sarà ad alto livello da parte del nostro Paese con i vertici dei Paesi più importanti e determinanti in questa battaglia.

(FLI). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il testo della mozione a prima firma della senatrice Bonino, il dibattito l'intervento del Governo mediante le parole e le riflessioni del sottosegretario Scotti, mi consentono di ribadire il parere favorevole del Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia attraverso una sola considerazione. Dalle parole del sottosegretario Scotti si evince che l'iniziativa parlamentare ha la possibilità di muoversi in due direzioni importanti. La prima lo è perché interviene nell'immediato su una questione che riguarda Tareq Aziz, cioè l'esigenza di consentire, come sottolineava il senatore Compagna,

di cui parlava il Sottosegretario, in direzione di un rafforzamento della tendenza a determinare condizioni internazionali per il superamento della pena di morte, dove ancora sussiste. quindi che l'iniziativa parlamentare oggi abbia questa duplice rilevanza: da una parte, dà un segnale di coralità del Parlamento e del Governo rispetto alla vicenda di Tareq Aziz; dall'altra, rafforza il percorso del nostro Paese, che sul terreno dei diritti civili deve muoversi con un orizzonte ed una forza ancora più significativi di quelli sinora manifestati. *(Applausi del senatore Saia).* Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Italia dei Valori vota in modo convinto a favore di questa mozione,

nella forza di una sottoscrizione internazionale, nell'impedimento all'accertamento della verità - un argomento che ha una notevole forza di persuasione - e, infine, nella necessità di essere coerenti con la moratoria internazionale stabilita dall'ONU il 18 dicembre 2007. A me pare meno rilevante il peso che parte significativa della stampa ha voluto dare sottolineando i caratteri della personalità dell'uomo,

Credo che questa condanna a morte, nelle condizioni storico-geografiche dell'Iraq, rappresenti a suo modo una sorta di illustrazione esplicita della qualità di quella che si vuole sia la democrazia irachena. Mi mordo subito la lingua, perché in realtà vi sono formidabili democrazie nel mondo che continuano ad usare questo stesso strumento. Indubbiamente, però, quel tipo di processo senza garanzie,

pena di morte. Credo che un'influenza, non solo nei confronti dell'Iraq ma anche degli Stati Uniti, circa l'uso della pena di morte potrebbe svolgere un ruolo importante a livello internazionale anche per convincere la

costringe noi occidentali a chiederci quale sia il nostro diritto di svolgere questa sorta di azione di maestri di democrazia. La condanna di Tareq Aziz è l'ultimo, l'ultimissimo atto di un processo che è cominciato con una guerra voluta a tutti i costi, basata su una colossale menzogna, sulla costruzione di una falsificazione di fatti, di cose e di intendimenti che parte proprio dall'Italia, perché il primo passo della falsificazione sulle armi di distruzione massa è partito dell'Italia. Questa guerra, voluta a tutti i costi, ha portato danni incalcolabili, stragi ripetute e abituali di civili coinvolti in bombardamenti e anche successive stragi nel corso Voglio inoltre ricordare, anche se qui può sembrare fuori posto, che la pratica distruttiva dell'intervento occidentale in Iraq ha prodotto altresì l'irrimediabile distruzione di un patrimonio culturale e artistico ultramillenario. Nella nostra memoria, penso in quella di tutti, nei nostri studi, il rogo della biblioteca di Alessandria sta come una sorta di *topos* della distruzione di cultura. Io vorrei che, con umiltà, quest'Aula e il Paese che sta fuori ricordassero ogni tanto che anche la biblioteca nazionale più importante di quel Paese è andata al rogo e che il museo più importante, che aveva al proprio interno una ricchezza culturale straordinaria, è stato dissipato da saccheggi e distruzioni.

democratico che dobbiamo portare dentro noi stessi: perché quel tipo di cose è accaduto, quel processo di distruzione è partito per un'iniziativa che noi abbiamo

luogo vorrei ringraziare lei, i radicali e Marco Pannella per questa iniziativa che abbiamo condiviso sottoscrivendo la mozione, perché

e persone che sono lontanissime da noi. Nel caso specifico, questa mozione è un atto dovuto, considerato che il Parlamento, non solo con riguardo alla moratoria sulla pena di morte, ma anche con la cancellazione - qualche anno fa - dell'ultima norma presente in Costituzione, relativa all'ammissibilità nell'ordinamento

della tutela della vita e della contrarietà alla pena di morte come strumento sanzionatorio. Quindi, credo che da questo punto di vista sia estremamente facile, soprattutto per noi, sostenere questa iniziativa. Essa però ha anche un sapore politico estremamente importante, perché serve a capire cosa sta succedendo in Iraq, come sta funzionando e se sta funzionando il progetto di ricostruzione sociale, civile, istituzionale, democratica, di quel Paese, se le condizioni in cui viene amministrata la giustizia in quel Paese obbediscono alle regole del diritto internazionale generalmente riconosciuto o se, viceversa, si tratta dell'esercizio di una ritorsione per ragioni religiose, per ragioni etniche, per ragioni varie. Certo, questa mozione non assolve Tareq Aziz né i suoi coimputati e non lo potrebbe fare. Questa mozione evidenzia che lui si è macchiato di crimini, come tutto *l'establishment* di Saddam Hussein, crimini determinati da condotte positive o omissive, ma che tutto ciò non giustifica la condanna a morte, la chiusura di chiusura di un'esperienza umana che determina peraltro, come molto opportunamente si dice nella nostra mozione, anche l'impossibilità di ricostruire quel periodo storico, le vicende che hanno riguardato i personaggi che ne sono stati protagonisti, le vere responsabilità: se non si ha, infatti, profonda conoscenza di tutto questo, in realtà non si può avviare a conclusione quel processo di democratizzazione di un Paese che, ancora oggi, versa in una condizione di criticità particolare. Aggiungo che a volte un atto di clemenza serve molto di più di tanti altri atti più o meno eclatanti, e che in questo caso, soprattutto dal punto di vista politico, interno ed esterno all'Iraq, un atto di clemenza che riguardi Tareq Aziz ed i suoi coimputati può servire ad avviare una fase nuova di riconciliazione reale in quel Paese che tanto ha bisogno non solo del nostro intervento, ma del nostro intervento a condizione che sia teso a farlo diventare totalmente un Paese civile. Queste sono le ragioni per le quali abbiamo convintamente

noi della Lega Nord, condividendone i contenuti del dispositivo e in considerazione della nostra ferma contrarietà alla pena capitale, voteremo convintamente in modo favorevole. Oggi il nostro però non è un no alla pena di morte per il criminale iracheno Aziz: vorrei sottolinearlo, oggi il nostro è un no fermo e deciso alla pena di morte. Nessuno, infatti, merita la morte, perché nessuno la può infliggere se non diventando, a sua volta, un omicida. Bisogna chiedersi: la pena capitale è effettivamente una vera e propria pena o, più semplicemente, un ulteriore delitto? La pena non va confusa con il concetto di vendetta. Tareq Aziz, come ogni delinquente, merita una pena, e in questo caso una pena sicuramente esemplare.

Se è vero che la pena è data a chi sbaglia per disincentivare gli errori e, quindi, per migliorare il mondo intero, allora uno Stato che commette un omicidio, a sua volta, non solo non migliora nulla in questo mondo, ma lo peggiora. Se è vero che una pena deve contenere anche un messaggio educativo e rieducativo, con la pena di morte muore anche il messaggio. Il Santo Padre ribadisce viva condanna della pena di morte, l'Unione europea sta intervenendo con forza per bloccare l'esecuzione il nostro ministro degli affari esteri Frattini ha già confermato l'appoggio dell'Italia alla richiesta di sospensione. Quindi, il no dell'Italia all'esecuzione arriva da ogni livello istituzionale. Dalla Cina il presidente della Repubblica Napolitano sostiene la posizione dell'Unione europea. Ma proprio la presenza a Pechino dovrebbe far assumere maggiore forza a questa denuncia, affinché sia una denuncia nei confronti di ogni condanna a morte, quindi anche di tutte quelle condanne a morte eseguite quotidianamente in Cina. Ricordiamolo, quindi. La Repubblica popolare cinese è uno dei Paesi in cui è applicata la pena di morte come sanzione ordinariamente prevista dal locale codice penale ed è il Paese con il maggior numero assoluto di esecuzioni capitali.

Come ricordava la signora Presidente, non si è persa neanche l'occasione per denunciare la condanna di Sakineh, ma dovrà essere sempre più forte il nostro impegno, affinché non nasca il sospetto che ci si muova a comando e solo per alcuni, magari qualcuno che è più famoso di altri. L'errore sarebbe ricordare l'orrore della pena capitale e l'inciviltà della condanna a morte solo in alcuni casi. Il sospetto che la comunità internazionale si muova ora solo perché Aziz, da Ministro degli esteri un tempo, come è stato ricordato in precedenza, è stato abile a crearsi amicizie internazionali, non deve essere nemmeno ipotizzabile, quantomeno da noi in quest'Aula. Aziz non va condannato a morte e non perché non lo meriti, ma perché nessuno può essere ucciso senza che venga a sua volta commesso un crimine.

una pena esemplare. Qualcuno a torto lo ha considerato il volto umano del regime iracheno; in realtà, è stato l'uomo più fedele di un dittatore criminale, Saddam Hussein. Ha ingannato tutti, provando a rappresentare la parte presentabile di una dittatura impresentabile. Da cristiano e cattolico incontrò il Papa, ma nulla ha fatto contro la nazionalizzazione delle scuole cristiane e l'insegnamento obbligatorio del Corano. Non solo: fu un attore della persecuzione e dell'eliminazione dei partiti religiosi in Iraq prima del 2003, della deportazione di popolazioni curde dalle regioni petrolifere del nord iracheno e delle esecuzioni a Baghdad del 1992. Difese anche anche Saddam in Aula, oltre che il sanguinario capo dei servizi segreti che considerava un fratello. Si presentava come un moderato in Occidente, ma poi nulla ha fatto per fermare i crimini del regime in patria. Nel 1980 fu proprio un fallito attentato ad Aziz a scatenare la guerra con l'Iran che in 10 anni provocò oltre un milione di morti. Non c'è dubbio Aziz sia un criminale e sia colpevole, ma un'esecuzione capitale aggiungerebbe soltanto un ulteriore crimine ai molti altri già compiuti. Ogni Paese civile sa che non potrà esserci giustizia commettendo un omicidio. Si faccia quindi giustizia vera e la si faccia proprio in un Paese come l'Iraq, che necessita di pace e che dovrebbe aver imparato ormai, come noi, che non può esserci vera pace senza giustizia.

all'ex ministro dell'interno Saadun Shaker e l'ex segretario personale di Saddam Hussein Abdel Hamid Hamud, è stato condannato a morte dall'Alta corte penale di Baghdad mediante impiccagione al termine di uno dei sette processi nei quali è imputato. Noi siamo coinvolti in questa vicenda per due ragioni fondamentali: ci sentiamo parte viva della comunità internazionale che, su nostra iniziativa, ha approvato il 18 dicembre 2007, nella sede dell'Assemblea dell'ONU, la moratoria universale della pena di morte, per la prima volta nella storia; la seconda, perché l'Occidente e noi con l'Occidente non siamo estranei al destino dell'Iraq. Oggi più di ieri siamo fortemente interessati a che l'Iraq diventi un grande Paese democratico, stabilizzato nella sua vita interna ed in grado di esercitare un ruolo di stabilizzazione dell'intera area. Sulla vendetta, signora Presidente, colleghi, non si costruisce nessuna democrazia; sulla vendetta delle vittime e sui carnefici, sulla ritorsione politica non si apre una stagione di pacifica convivenza. Lo sanno bene i Paesi - e l'Italia è tra questi - che hanno dovuto ricostruirsi dopo tragedie devastanti, violenze ed uccisioni. La ricostruzione, per essere solida e duratura, non può che fondarsi sul riconoscimento delle responsabilità e delle sofferenze reciproche e su una scelta condivisa, sul valore della vita, della persona e dei diritti umani, valori assoluti. La persona e la storia: uno dei temi cruciali della storia del XXI secolo sotto tutti i cieli perché appunto la storia di tanti secoli ci ha consegnato questa sfida. Un destino comune si assicura così perché solo così la generazione che è coinvolta in questo passaggio può consegnare alle nuove generazioni un patrimonio di verità e di fiducia, con una storica discontinuità, con gli errori e le colpe dei padri. Non è la stessa cosa consegnare alle nuove generazioni la memoria della vendetta o della verità, della clemenza, della riconciliazione. Solo quest'ultima memoria è feconda per il futuro. Noi siamo coinvolti nel destino dell'Iraq anche perché siamo stati attori, assieme all'Occidente, di quella guerra che noi continuiamo a considerare un errore storico e politico, le cui conseguenze oggi ci interpellano perché è proprio in ragione di quelle responsabilità che noi oggi siamo fortemente impegnati a difendere con tutte le nostre forze il diritto internazionale che appunto ha fissato standard di giustizia che escludono la pena di morte. Ed è sulla base di questo nostro legame con l'Iraq che il sangue versato dai militari e civili italiani ha fortificato, che oggi noi diciamo a quel Paese: non ripetete gli errori del passato, interrompete la catena di violenze, di crimini e di violazioni dei diritti umani che Saddam ha avviato. Riconosciamo insieme che solo il diritto internazionale è la bussola del nostro futuro comune. Un altro pensiero motiva la nostra azione perché sia evitata l'esecuzione di Tareq Aziz e degli altri coimputati. Essi sono stati protagonisti del regime di Saddam Hussein e delle sue scelte, e perciò ne sono anche testimoni. Sono in un certo senso due profili che vanno colti con distinzione: sono gli ultimi testimoni, non si possono distruggere. Bisogna sapere che, quando si è di fronte a tragedie politiche di questa portata,

In un certo senso, la cancellazione dei testimoni non è nelle disponibilità del potere. Lo stesso accertamento della verità su tutta la vicenda dell'Iraq, che ci ha coinvolto, è un dovere anche per noi, noi, come si è detto, anche attraverso la Commissione d'inchiesta. Anche per noi la verità è una struttura decisiva per la democrazia. Non ripetere gli errori è uno dei vantaggi della democrazia. Signora Presidente, la mozione che abbiamo presentato esprime per il nostro tramite la volontà del popolo italiano di sviluppare il suo rapporto di collaborazione con il popolo iracheno, sulla base di grandi valori condivisi. Un rapporto che ha origini antiche: da Ur dei Caldei partì Abramo, il comune padre delle tre grandi religioni monoteiste, l'ebraica, la cristiana, la musulmana. un rapporto che ha visto la presenza dei nostri connazionali nella vita economica, civile e culturale dell'Iraq prima della guerra, nella stessa costruzione della precedente città di Baghdad e nella sua urbanistica, che vede anche oggi la realizzazione di progetti di ricostruzione materiale, sociale e culturale con presenza italiana. Chiediamo, dunque, che il nostro Governo si faccia interprete di questa unanime volontà, così come il sottosegretario Scotti ha di recente dichiarato, adoperandosi in tutte le sedi perché sia evitata l'esecuzione di Tareq Aziz e dei suoi coimputati e perché l'Unione europea faccia formale richiesta alle autorità irachene di reintrodurre la moratoria della pena di morte, stabilita in Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein, come pilastro essenziale per il completamento della transizione democratica.

Per queste ragioni, l'Europa è amata nel mondo. In questi giorni Marco Pannella ha ripreso il suo *satyagraha*, rendendosi quasi simbolo esistenziale di una richiesta che è tra le più alte che l'umanità e una matura coscienza politica possano esprimere. Il Gruppo del Partito Democratico guarda al futuro democratico dell'Iraq con fiducia e speranza. Si sente fortemente vicino al popolo iracheno e con franchezza si rivolge al suo Governo e ai suoi rappresentanti perché facciano dell'Iraq un Paese che in tutta l'area del Medio Oriente, alle porte dell'Asia, apra la strada alla riconciliazione, alla democrazia, ai diritti umani, alla pace. Vivono questi sentimenti e questa volontà nel voto favorevole alla mozione che il Gruppo esprimerà; ma vive anche la memoria che nelle vicende dei popoli solo l'affermazione del diritto, della verità, del rispetto della vita possono assicurare (e lo possono assicurare solo insieme) un futuro di prosperità. È nel cuore di questa visione che l'esecuzione della condanna di Tareq Aziz e dei coimputati può e deve essere evitata.

*(PdL)*. Signora Presidente, vista la tarda ora leggerò soltanto alcuni passaggi della dichiarazione di voto a nome del Popolo della Libertà, consegnando poi il testo direttamente agli Uffici. colleghi, con la mozione oggi al nostro esame abbiamo voluto riproporre in quest'Aula, prima e ancor più che una questione particolare, un tema generale. Vogliamo riaffermare un valore profondo in cui crediamo e un impegno, quello di abolire la pena di morte in qualsiasi circostanza, al quale ci sentiamo moralmente e politicamente legati. Un impegno cui la nostra legislazione già da tempo è perfettamente allineata, da ultimo con l'approvazione, proprio all'inizio di questa legislatura, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che afferma e perfeziona quel diritto comune europeo che fa del nostro continente uno spazio di diritti esenti dalla pena di morte. È un principio che abbiamo voluto iscrivere nei documenti fondanti l'identità della nostra unione, l'Unione europea, a partire dalla Carta dei diritti fondamentali. Credo che, volgendoci alla nostra storia, noi italiani dobbiamo rivendicare con orgoglio il contributo dato alla costruzione di questo diritto comune europeo. Ricordo che nel 1786, nella mia Toscana, fu per la prima volta abolita la pena di morte in Europa e che è - chi per primo fornì in modo compiuto gli argomenti per rovesciare una tradizione europea di legislazioni fondate sulla pena di monte e sulla sua legittimità. Forti di questa tradizione, abbiamo saputo, sulla base del continuo stimolo che proveniva dalle forze politiche e dalla nostra società civile, portare questa battaglia a livello internazionale. Sono queste ragioni, le stesse che motivano la nostra battaglia a livello internazionale, a spingerci oggi a chiedere di evitare l'esecuzione di Tareq Aziz. Chiedere la sospensione di questa pena vuole testimoniare una volta di più il nostro impegno per la moratoria universale della pena di monte. Non posso non ricordare i miei incontri con Tareq Aziz, fino all'ultimo, all'immediata vigilia dello scoppio della guerra in Iraq; un uomo, certo, responsabile ai più alti livelli delle scelte del regime, ma sempre orientato a cercare comprensione e soluzioni. Sono convinto che per l'Iraq ribadire la scelta già fatta a suo tempo di sospendere l'esecuzione di questa e di tutte le pene capitali sia la migliore testimonianza dei progressi di uno Stato che vuole essere perfettamente inserito nella comunità internazionale. In una Nazione che ha recuperato la sua libertà, che ha superato l'anarchia, che vede, come diceva Beccaria, il regno delle leggi, dov'è la necessità di distruggere un cittadino? Sarà la sua morte il freno per distogliere gli altri dal commettere delitti o, in quella tormentata parte del mondo, non sarà piuttosto il segno di una società divisa, che non sa fare pace con la storia? Con queste convinzioni, nel dichiarare il voto favorevole del Popolo della Libertà alla mozione, credo che il Parlamento italiano si debba unire alla richiesta che viene dalle più alte istanze dell'Unione europea di una moratoria dell'esecuzione di una pena crudele e inumana, che rappresenta un inaccettabile diniego della dignità dell'uomo e della sua integrità.

dire qui che condivido le ragioni politiche, morali e giuridiche con le quali si chiede la sospensione dell'esecuzione della pena di morte di Tareq Aziz e delle altre persone con lui condannate. Desidero anche esprimere la mia condivisione delle ragioni con le quali si riafferma qui la richiesta della moratoria della pena capitale. Aggiungo che a questa mia dichiarazione di voto non sono estranei il rapporto intrattenuto in tempi andati con Tareq Aziz, ancor prima del Kuwait da parte di Baghdad, e le ragioni di rispetto personale che ho maturato in quelle circostanze. Aggiungo, infine, la mia richiesta

Egregia Presidente, colleghi senatori, desidero in qualche modo rendere ragione, con questo breve intervento, del mio voto di astensione, e quindi in difformità rispetto alle scelte tanto del partito di appartenenza, quanto dello stesso Governo. Una posizione, la mia, che discende dal convincimento di una funzione, comunque, positiva, anche sotto il profilo della giustizia intesa come *ius*, come diritto, della pena di morte. Si diceva un tempo, in ambito rigorosamente cattolico, che due erano le giustificazioni per questa forma estrema di condanna: «*quia peccatum est*», nel senso che, di fronte a reati particolarmente efferati, non vi poteva essere un'altra risposta, non c'era una risposta corrispondente e adeguata, e «*ne peccetur*», perché, comunque, la pena di morte rappresenta un deterrente sicuramente significativo. un dubbio, soprattutto in relazione alla possibile applicazione della pena di morte in una realtà come quella italiana, con una magistratura che in alcune componenti soffre di due forme endemiche di malattia.

della loro funzione, uno stile di vita. Non avevano bisogno, come in Inghilterra, della parrucca: diverso era il loro comportamento. soffermare l'attenzione su un altro aspetto che mi sembra particolare e addirittura emblematico di uno stato di confusione e di una perdita di riferimenti. È passata una certa filosofia tutta di sinistra

il proliferare e i finanziamenti continui ad associazioni che si interessano in forma esclusiva di detenuti. Nella mia sola provincia vengono tenuti corsi di danza, di recitazione, di essenze e profumi, di pari opportunità

Vorrei ricordare Giovannino Guareschi, un grandissimo italiano che, quando all'uscita dal carcere di Parma venne intervistato dai giornalisti che gli chiedevano con insistenza se all'interno del carcere avesse trovato persone che pativano ingiustamente privazioni per quello stato e per quelle condizioni, rispose, con l'ironia che gli era tipica: sì, moltissimi, tutti gli agenti di custodia. Non entro poi nel merito della questione specifica

delle forme di repressione più estreme, quindi non ho elementi di valutazione. Posso fare una considerazione: quando ci sono i processi dei vincitori sui vinti, è difficile che vi siano equilibrio e giustizia.

capire che fine ha fatto il disegno di legge Alfano, impropriamente chiamato svuota-carceri, ma più testualmente titolato: «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno».

per lo meno si prevedeva la possibile assunzione di 2.000 agenti penitenziari, e ciò avrebbe potuto comportare l'apertura di alcuni reparti, e quindi avrebbe consentito di intervenire sul sovraffollamento penitenziario.

55 sono i suicidi dall'inizio dell'anno), forse è il caso che lo stesso Governo si prenda un impegno sull'*iter* di questo intervento legislativo che, seppur minimale, rappresenta un segnale per il nostro sistema penitenziario.

Auspico, quindi, che venga colmata da parte del Governo tale gravissima inadempienza, che non può continuare. Inoltre, signora Presidente, approfitto per sollecitare la